L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

formale, vorrei soltanto dire che poco fa sono passato a trovare il presidente emerito Giorgio Napolitano, che mi ha chiesto di salutare tutti i membri dell'Assemblea.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il mio intervento di oggi intende rendervi partecipi degli argomenti in discussione nel Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di un passaggio importante e vi ringrazio di essere qui. L'interlocuzione con il Parlamento è essenziale per definire la posizione del nostro Paese su temi di grande rilevanza per la vita dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni. Procederò a toccare i principali temi in agenda, che includono la ripresa economica, la pandemia da Covid-19, i vaccini, le migrazioni, temi di politica estera, come i rapporti con Turchia e Russia, e le crisi in Etiopia e nel Sahel. La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2 e del 4,4 cento, come il resto dell'Unione europea nel suo complesso. Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione indicano però che la ripresa sarà ancora più sostenuta. Gli ultimi dati sulla fiducia di imprese e consumatori, riferiti al mese di maggio, sono in marcato aumento. Il dato per le imprese, in particolare, è in forte accelerazione rispetto alla tendenza positiva degli ultimi mesi ed è il dato più alto dal febbraio 2018. Anche il commercio estero è ripartito. Nel mese di aprile, le esportazioni sono cresciute notevolmente, non solo rispetto all'anno scorso, quando il loro livello era stato eccezionalmente basso, ma anche rispetto a due anni fa, segnando un aumento del 7,4 per cento. Sempre ad aprile, l'indice della produzione industriale è aumentato dell'1,8 per cento rispetto a marzo. La fiducia, insomma, sta tornando. Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile i tassi di crescita anemici che l'Italia registrava prima della pandemia. Per far ciò è fondamentale mantenere a livello europeo una politica di bilancio espansiva nei prossimi mesi. Durante la pandemia abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della nostra economia, ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta. Abbiamo protetto l'offerta durante la pandemia, mantenuto e protetto i posti di lavoro e l'occupazione e aiutato le imprese a superare le situazione di crisi di liquidità: ora dobbiamo mantenere alta la domanda, al livello di tale offerta. Raggiungere tassi di crescita notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni ci permetterà anche di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che è aumentato di molto durante la pandemia, e ci consentirà di creare nuovi lavori, fondamentali per affrontare le transizioni, come quella digitale e quella ambientale. In questo quadro economico positivo permangono, però, alcuni rischi. Il primo è proprio la situazione epidemiologica, di cui parlerò più avanti nel mio intervento. Sebbene in forte miglioramento, questa dev'essere osservata e monitorata con molta attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l'emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti. Il secondo potenziale pericolo è l'inflazione che, nell'area dell'euro, ha raggiunto il 2 per cento a maggio, dopo l'1,6 per C'è largo consenso che, a oggi, questo aumento sia temporaneo, perché legato a un recupero della domanda, a strozzature dell'offerta e a effetti contabili. L'inflazione cosiddetta *core* - che esclude le componenti più variabili, come l'energia - rimane molto bassa nella zona

Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, affinché le aspettative di inflazione restino ancorate all'obiettivo di medio termine. Dobbiamo guardare anche al rischio di una divergenza tra l'economia della zona euro e quella statunitense e le implicazioni che essa potrebbe avere per la politica monetaria della Federal reserve e della Banca centrale europea. Un ulteriore rischio è legato al debito. Nel corso del 2020 il rapporto debito-PIL nell'Unione europea è salito di 16,7 punti percentuali, in Spagna di 25,7, in Francia di 18,5 e in Italia di 15,8 punti. Nel 2020 i Governi europei hanno utilizzato in maniera corposa le garanzie statali per un totale di 450 miliardi di euro nei soli quattro Paesi più grandi dell'Unione. È prevedibile che parte di queste garanzie sarà dovuta e quindi provocheranno un ulteriore aumento di debito. Tuttavia, una politica di bilancio espansiva rimane essenziale per preservare ritmi di crescita sostenuti che, a loro volta, permetteranno di ridurre l'indebitamento. È però importante che tutti Governi si impegnino a tornare a una politica di bilancio prudente, nel medio e anche lungo termine, una volta che la crescita sarà di nuovo sostenibile. Ciò serve a rassicurare gli investitori e i mercati, a prevenire eventuali rialzi dei tassi di interesse e dunque favorire gli attuali programmi di investimento. L'ultimo rischio riguarda la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa dalle crisi recenti hanno spesso favorito solo alcune fasce della popolazione, penalizzando i meno abbienti, i più giovani e le donne. Non abbiamo prestato la dovuta attenzione alla crisi climatica che colpisce soprattutto le aree più fragili del Paese. Questa volta dobbiamo e vogliamo agire diversamente. Ad esempio, dobbiamo mettere in campo politiche attive del lavoro efficaci per aiutare chi ha bisogno di formazione per trovare un nuovo impiego. Il Consiglio europeo discuterà di come garantire una crescita durevole e sostenibile anche grazie alle risorse del Next generation EU. A livello europeo è molto positivo che 24 dei 27 piani dei Paesi membri siano già stati formalmente presentati e che la Commissione ne abbia già esaminati L'erogazione dei fondi dipenderà dall'approvazione da parte del Consiglio ed è importante che questo avvenga in modo rapido ed efficace. L'approvazione del Piano italiano da parte della Commissione, confermata dalla presidente von der Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, attesta il grande lavoro svolto dal nostro Paese. Abbiamo messo insieme un piano ambizioso di riforme e investimenti e lo abbiamo fatto con la collaborazione degli enti territoriali, delle parti sociali e del Parlamento, che tengo qui a ringraziare. Il vostro ruolo come Parlamento continuerà a essere fondamentale durante tutta l'attuazione del piano. Come ho avuto modo di dire ieri alla presidente von der Leyen, l'approvazione da parte della Commissione è solo il primo passo. Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo per avviare i progetti di investimento previsti e portare avanti l'agenda di riforme. Gli occhi dell'Europa sono sull'Italia, su di noi. Il nostro è infatti il programma più significativo e sostanzioso, per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare. Il successo del programma Next generation EU dipende solo da noi. Per quanto riguarda la pandemia, rispetto alle mie comunicazioni alle Camere del 24 marzo scorso, il quadro epidemiologico in Italia - e in generale in Europa - è molto migliorato. La scorsa settimana in tutta l'Unione europea abbiamo registrato circa 90.000 casi e ci sono stati 2.600 decessi dovuti al Covid-19. Due mesi fa i casi erano circa un milione a settimana e i decessi settimanali sei volte quelli attuali. Questo miglioramento è merito della campagna vaccinale, che procede in maniera spedita. A metà aprile in Italia solo un adulto su quattro aveva ricevuto almeno una dose e appena uno su dieci aveva completato il ciclo vaccinale. A oggi, nell'Unione europea più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino. In Italia la quota è pari a e circa il 30 per cento della popolazione adulta ha completato l'intero ciclo di vaccinazione. I rischi legati alle varianti, e in particolare alla cosiddetta variante Delta, ci impongono di procedere nella campagna vaccinale con la massima intensità. Dobbiamo inoltre continuare a concentrarci sui soggetti più fragili, come i più anziani, che sono maggiormente a rischio di morte o di ospedalizzazione. La priorità è cercare tutti gli *over* 50 ovunque essi siano e vaccinare, oppure cercare di persuadere quelli che non vogliono avvicinarsi, ma questa è la priorità assoluta, oggi, della campagna di vaccinazione. Per quanto riguarda il *pass* italiano, il 17 giugno è stato firmato il DPCM che definisce le modalità di rilascio e poco fa il ministro Speranza mi ha comunicato che in più di cinque milioni hanno già scaricato il certificato di vaccinazione. È quindi operativa in Italia la piattaforma informatica di rilascio della certificazione, che facilita la partecipazione ad alcune tipologie di eventi e gli spostamenti tra Regioni in caso di peggioramento del quadro epidemiologico. Dal 1° luglio la certificazione sarà valida anche come certificato verde europeo per poter viaggiare da e per i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Intanto consentiamo già, alle stesse condizioni di certificazione, l'ingresso in Italia dei turisti provenienti dalle stesse aree, dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Giappone; insomma, vogliamo permettere loro di venire in sicurezza in Italia, per aiutare i nostri albergatori, il turismo e i ristoratori a ripartire, dopo un anno e mezzo di difficoltà. Sempre sul tema dei vaccini, il Consiglio europeo affronterà nuovamente la questione della solidarietà internazionale: migliorare l'accesso ai vaccini nei Paesi più poveri non è soltanto una questione etica, ma anche una priorità sanitaria. Più a lungo dura la pandemia, più possibilità ci sono che il virus muti in varianti particolarmente contagiose, che possono sfuggire alla copertura del vaccino. Anche su questo fronte sono stati fatti importanti passi in avanti nel corso degli ultimi due mesi. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto al Global health summit organizzato dall'Italia insieme alla Commissione europea, a Roma, il 21 maggio scorso. Il *summit* è stato il preludio del Consiglio europeo straordinario del 24-25 maggio, in cui i Paesi dell'Unione europea si sono impegnati a donare almeno 100 milioni di dosi di vaccini entro la fine dell'anno. L'Italia farà la sua parte e donerà 15 milioni di dosi quest'anno. Nel vertice G7 in Cornovaglia e nel successivo vertice Unione europea-Stati Uniti, è stato ribadito l'impegno comune ad aumentare la produzione dei vaccini anche al fine di una loro distribuzione più equa a livello globale. Come ho dichiarato in altre occasioni, il trasferimento di tecnologie verso Paesi terzi è molto utile a questo fine; tale questione andrà definita nel quadro di un negoziato presso l'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione è pronta a presentare una propria proposta scritta come base per i negoziati. Al Global health summit la presidente von der Leyen ha presentato l'iniziativa europea per la produzione locale e l'accesso ai vaccini, ai farmaci e alle tecnologie sanitarie nel continente africano; è un'iniziativa che l'Italia appoggia con determinazione e convinzione. È previsto un miliardo di euro in investimenti a carico del bilancio europeo da incrementare col supporto degli Stati membri. il Consiglio europeo verrà inoltre accolta la decisione, adottata dalla settantaquattresima Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, di convocare una sessione speciale dell'Assemblea mondiale della salute a novembre. In quell'occasione si discuterà di un quadro comune per migliorare la preparazione globale a future pandemie sulla base delle lezioni apprese durante questa crisi sanitaria. L'Italia, come tanti altri Paesi, si è trovata impreparata all'arrivo Non possiamo e non vogliamo permettere che questo accada di nuovo. La Dichiarazione di Roma, approvata anch'essa al Global health summit, fornisce un'ottima base per una maggiore cooperazione e solidarietà internazionale in futuro. Un altro tema che ci riguarda da vicino è la gestione dei flussi migratori, che torna a essere in agenda del Consiglio europeo su precisa richiesta dell'Italia. Pensate che non era più nell'agenda del Consiglio europeo dal giugno 2018. Come ho dichiarato in passato, il Governo vuole gestire l'immigrazione in modo equilibrato, efficace e umano, ma questa gestione non può essere soltanto italiana; dev'essere davvero europea. Occorre un impegno comune, che serva a contenere i flussi di immigrazione illegali, a organizzare l'immigrazione legale e aiutare questi Paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace (e penso ovviamente, in modo particolare, alla Libia). Un miglior controllo della frontiera esterna dell'Unione può essere la base per un piano più ampio, che comprenda anche il tema dei ricollocamenti. Tra i Paesi dell'Unione esiste un'ampia convergenza sull'esigenza di superare il Regolamento di Dublino. Si tratta di una convenzione concepita in una diversa fase storica, adatta a gestire numeri contenuti. Al momento, però, una solidarietà obbligatoria verso i Paesi di primo arrivo, attraverso la presa in carico dei salvati in mare, rimane divisiva per i 27 Stati membri. Serve un'alternativa di lungo periodo, per fare in modo che nessun Paese sia lasciato solo. Il Patto sulla migrazione e l'asilo, proposto il 23 settembre dello scorso anno dalla Commissione europea, ha il merito di ricercare un cambio di prospettiva. Il negoziato sul Patto dimostra, tuttavia, che c'è ancora molto lavoro da fare. Attualmente sta emergendo un terreno comune fra gli Stati europei su diversi aspetti fondamentali. Tra i 27 Stati membri ci sono punti di convergenza, innanzitutto sul riconoscimento delle rotte migratorie come parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea. Intendiamo intensificare in tempi rapidi partenariati e forme di collaborazione con i Paesi di origine e di transito, in particolare con quelli africani. Lo scopo è evitare perdite di vite umane, ma anche contrastare le partenze illegali, nonché ridurre la pressione sui confini europei. *(Applausi)*. Ho discusso anche di questo durante gli incontri avvenuti nelle ultime settimane con il primo ministro libico Dabaiba e il presidente della Repubblica tunisina Saïed, dai quali ho ricevuto riscontri positivi. Anche la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito l'urgenza di portare avanti azioni concrete dai tempi certi con i Paesi di origine e di transito, un invito su cui mi sembra ci sia ampia convergenza. Inoltre, la maggioranza dei Paesi membri sembra essere sensibile all'esigenza di una più stretta collaborazione tra l'Unione europea, l'Alto commissariato ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni riguardo a tutte le rotte migratorie. Vogliamo che il Consiglio promuova un'azione più incisiva sui rimpatri, anche attraverso lo strumento dei rimpatri volontari assistiti, e che favorisca un impegno comune a sostegno dei corridoi umanitari. Credo che finora siamo solo noi che riusciamo a farlo. Lo facciamo anche abbastanza bene, ma chiaramente sono numeri abbastanza piccoli. Più in generale, serve una maggiore considerazione dal punto di vista politico e finanziario delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale e occidentale. Oggi è privilegiata dall'Unione europea soprattutto la rotta orientale sul piano giuridico e finanziario. Occorre uno specifico impegno dell'Unione europea per la stabilità in Libia, auspicabilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la politica estera, il Consiglio europeo si occuperà prima di tutto dei rapporti tra Unione europea e Turchia. Nella sua riunione di marzo, il Consiglio aveva ricordato come sia di interesse strategico europeo avere una situazione di stabilità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e dunque collaborare con la Turchia. Il Consiglio intende sottolineare di nuovo la disponibilità dell'Unione europea a cooperare in alcune aree di interesse comune, come la lotta ai cambiamenti climatici, la salute pubblica o la lotta al terrorismo. Siamo impegnati anche sul tema dell'unione doganale. Ribadiremo però la nostra preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, come i diritti delle donne, i diritti civili e i diritti umani. Per quanto riguarda la Russia, si farà riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di maggio e si ribadirà l'impegno ai principi chiave che governano la relazione tra Unione europea e Russia. Infine, nelle conclusioni del Consiglio europeo sono previsti riferimenti alle crisi nel Sahel e in Etiopia. La stabilizzazione del Sahel rappresenta una priorità per l'Italia. Negli ultimi anni abbiamo ampliato il nostro impegno nella regione sia sul piano politico, sia su quello della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza nel campo della sicurezza. A riprova dell'attenzione italiana ed europea alla stabilità nella regione del Sahel, è opportuno ricordare la nomina, il 21 giugno, dell'onorevole Emanuela Claudia Del Re come rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel. Per quanto riguarda la grave crisi umanitaria nel Tigrai, l'Italia continua a fare appello per un immediato cessate il fuoco, il pieno accesso umanitario e la fine degli spostamenti forzati. Chiediamo inoltre indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e l'avvio di un percorso di riconciliazione nazionale. Lo facciamo nel solco dei tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione bilaterale e nel pieno sostegno al processo di riforme e allo sviluppo del Paese.

la campagna vaccinale ci sta permettendo di contenere in maniera efficace la pandemia, la ripresa economica procede rapida e il programma Next generation EU ci fa guardare con fiducia a una stagione di riforme e investimenti. Tuttavia, permangono diverse sfide, a partire dalla gestione della migrazione, che dobbiamo affrontare con attenzione per andare incontro alle richieste dei nostri cittadini. L'Unione europea è la sede giusta per risolvere questi problemi, ma è importante che i nostri *partner* comprendano l'urgenza di trovare soluzioni rapide e condivise. Il vostro sostegno è e sarà determinante per portare avanti gli interessi italiani in Europa.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

Signor Presidente, l'ultima esperienza che ho avuto parlando in quest'Aula, nella quale sono stato interrotto dopo dieci minuti - non certamente per responsabilità di alcuno, salvo che del Regolamento - mi induce a essere sintetico e annunciarle che vorrei parlare di tre cose. Vorrei parlare del suo discorso, di lei e di noi. Vorrei parlare del suo discorso, del professor Draghi e di noi parlamentari.

c'è una prospettiva incoraggiante dell'economia, non sottovalutando i rischi che incontreremo alla ripresa autunnale. Le vaccinazioni vanno bene, vanno meglio, e il tema dell'immigrazione, come sa bene la Ministra dell'interno, è un'autentica emergenza, ma purtroppo siamo soli. Lo ha ricordato anche lei,

tutti noi la accompagniamo al Consiglio europeo con assoluta e convinta solidarietà. Adesso parliamo di Draghi e parliamo di noi. Vorrei farlo senza adulazione, peraltro assai in voga in questo periodo, e senza ipocrisia, sempre in voga nella politica. Come è capitato in tanti momenti della vita nazionale, siamo andati a cercare un signore di grande prestigio, non eletto in Parlamento - era infatti fuori dal Parlamento perché ci trovavamo in una condizione di assoluta emergenza. Lo abbiamo fatto e il professor Draghi ha accettato di mettere non solo la sua capacità tecnico-politica, ma anche e soprattutto il suo nome, come ombrello protettivo di un Paese...

se è vero che è un ombrello efficacissimo e un efficacissimo interprete della politica italiana rispetto ai temi del *recovery* *plan* e del rapporto con l'Europa, noi dobbiamo avere - qui parlo di noi - l'onestà intellettuale di capire che i problemi sono esattamente gli stessi e sono tutti davanti a noi.

non è una battuta, ma l'indicazione preoccupante di una marginalità crescente, che il Parlamento deve registrare. Se non ci rendiamo conto di questo,

attendere e metterci in una situazione di paralisi e di attesa, rispetto alla questione delle riforme e degli investimenti che sono necessari, oppure affrontare i problemi.

In primo luogo, il professor Draghi ha parlato di competitività anemica - credo che abbia usato giustamente questo termine - italiana, per cui cresciamo meno degli altri Paesi, crescevamo meno anche prima e dobbiamo crescere di più, se vogliamo non solo utilizzare i soldi del *recovery* *plan*, ma utilizzare l'occasione che dalla pandemia ci viene offerta. questioni da affrontare non c'è solo quella della pubblica amministrazione, ma anche quella della giustizia. Vorrei dire una cosa con molta semplicità e chiarezza: i provvedimenti sulla giustizia non possono essere un pannicello caldo. Non servono i pannicelli caldi, perché oggi abbiamo questioni emergenziali. Basta pensare al livello di discredito che nell'opinione pubblica hanno i magistrati e confrontarlo con il rispetto assoluto reputazionale che avevano vent'anni fa. Ebbene, colleghi, non basta una riforma del CSM, che, peraltro, dilata il numero dei componenti del CSM stesso (questo, francamente, è un po' sorprendente), senza una separazione netta tra le sezioni disciplinari e l'organo amministrativo. Sulle valutazioni professionali dei magistrati verrebbero introdotti altri indici e altri parametri, che, come sappiamo tutti, aumenteranno il contenzioso al TAR: perché chiunque oggi viene bocciato in una sede in cui vorrebbe andare, unica azione immediata il ricorso al TAR. E il contenzioso amministrativo aumenta. Ci vuole il coraggio di dire che, se un pubblico ministero manda a processo centinaia di persone che regolarmente vengono assolte, questo, in termini di valutazione professionale, non può che essere una cosa discreditante, perché in un'azienda privata tutti adotterebbero questo sistema.

noi abbiamo introdotto sulla vostra spinta. Molti Paesi hanno un reddito di cittadinanza, sotto forme diverse. Benissimo: credo sia importante dare una tutela alle fasce emarginate, ma attenzione: si stanno moltiplicando gli episodi di datori di lavoro che, forse anche a causa di regole non chiarite,

In Libia siamo in una situazione emergenziale assoluta e in una condizione in cui non abbiamo carte da dare. io capisco di affrontare un altro tabù, ma ci rendiamo conto di essere gli unici *player* mediterranei che sono riusciti a litigare, nello stesso momento, con l'Egitto e con la Turchia,

noi come Parlamento e poi successivamente il Governo, un esame serio. Abbiamo dei contenziosi che vanno affrontati. Sono dolorosi, riguardano vicende umane e quei quei diritti dell'uomo cui, giustamente, il presidente Draghi ha fatto riferimento. Sono orgoglioso che il mio Presidente del Consiglio faccia tali affermazioni, perché sono la storia e la tradizione italiana, ma, colleghi, noi dobbiamo mirare a cambiare una politica che, se non ci dà la possibilità di essere punto di riferimento nel Mediterraneo, ci condanna ad una subalternità permanente. Erano le questioni che voleva affrontare. Credo e spero siano state di qualche utilità.

Presidente del Consiglio, l'incontro di ieri tra lei e la presidente *von der Leyen* offre l'occasione migliore e rende doveroso e gradito rallegrarci con lei, per la sua *leadership* in Italia, in Europa ed oltre l'Europa, e rallegrarci con l'Unione europea per la risposta, che è stata, contemporaneamente, visionaria ed estremamente concreta alla crisi pandemica. Tocco rapidamente due punti. Il primo è brevissimo ed è di particolare apprezzamento per il modo in cui lei, presidente Draghi, ha descritto le prospettive del quadro economico, un modo particolarmente equilibrato, senza alcun allarme per ora, ma menzionando i temi dell'inflazione e del debito che, senza alcuna soverchia preoccupazione oggi, meritano però grande attenzione. La mia seconda osservazione è sull'Europa. Lei ci ha mostrato, anche con l'evento di ieri sul PNRR, l'Europa che funziona e funziona bene, ci ha mostrato, con i suoi riferimenti all'agenda del Consiglio europeo al quale si accinge a partecipare, anche l'Europa che per ora non funziona:

un accordo sulla tassazione minima delle società; le vere difficoltà saranno poi in Europa per farla approvare da tutti gli Stati membri. membri. Lei ha invocato soluzioni rapide e condivise. In questi tre campi i progressi sono insufficienti, faticosi e lenti. La radice comune a questi tre e ad altri punti di difficoltà dell'Unione europea, come lei sa bene, è che in queste materie non può decidere, se non con il vincolo dell'unanimità. La mia domanda è di prospettiva: nella prospettiva della Conferenza sul futuro dell'Europa, le chiedo come il Presidente del Consiglio italiano la possibilità, la strategia e le modalità per andare gradualmente, se lo ritiene necessario, verso superamenti, almeno parziali e condizionati,

Presidente Draghi, mi permetta di dirle grazie. Grazie per il lavoro che sta portando avanti con autorevolezza e competenza, che di rimando sono attribuite nuovamente - e direi finalmente - anche al nostro Paese. Risulta ovvio, almeno dal mio punto di vista, che c'è stato un netto cambiamento in Europa rispetto al passato. È sotto gli occhi di tutti quanto lei sia rispettato dagli altri *leader* europei, quanto le posizioni dell'Italia abbiano una voce forte e quanto in questi mesi sia decisamente cambiato il passo, non solo nella gestione della pandemia e della fase economica, ma proprio nei rapporti con tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea. Il prossimo Consiglio europeo sentirà forte le posizioni dell'Italia sui temi importanti che lei ha ben focalizzato e ricordato con nettezza e chiarezza. Proprio perché è stato netto e chiaro, soprattutto sul piano economico e pandemico, non mi sento assolutamente, né di ritornare sui soliti argomenti, né di darle consigli, che mi pare del tutto evidente non sono necessari. Mi prendo quindi la libertà di spostare l'attenzione su altre tematiche che lei ha toccato, anche alla luce degli eventi di cronaca politica dell'ultimo periodo. Nel suo discorso ha parlato di Europa a 360 gradi, ha parlato di economia e ha fatto capire come il PNRR non sia un regalo, ma una risposta alle oggettive difficoltà economiche che l'Italia ha affrontato e continua ad affrontare. Ha parlato di pandemia, ma ha anche affrontato il tema fondamentale della transizione digitale e anche per questo la ringrazio, perché il futuro di un Paese non può prescindere dalla sua digitalizzazione. Stesso discorso vale per la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale, entrambi argomenti di chi guarda al futuro del Paese a lungo raggio. Lei ha poi parlato di Turchia, di Libia, di flussi migratori, di ripresa dei rapporti internazionali. Tutto questo di rimando non può che portare anche ad una riflessione legata al rapporto che l'Europa ha con i diritti. Anche se l'Unione europea è l'area del mondo che assicura la maggiore tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, negli ultimi tempi vi sono stati degli arretramenti o addirittura delle chiare violazioni sulle libertà personali, sui diritti delle minoranze e sulla libertà di accesso alla libera informazione, arretramenti su cui l'Unione europea non può tacere senza minare il proprio progresso sociale e culturale. Se parliamo di immigrazione, ad esempio, non possiamo tralasciare la situazione gravissima che sta affrontando la rotta orientale sin dal 2017. Con lei, presidente Draghi, l'immigrazione è tornata al centro dei dibattiti europei per cercare di ottenere, come lei ha detto, una soluzione equilibrata, efficace, ma soprattutto umana. La sua onestà intellettuale le fa parlare di immigrazione associata a una necessaria integrazione, unico connubio possibile per una gestione concreta e adeguata del problema. Forza Italia non può che accogliere con favore la ripresa dei contatti tra Italia e Libia. I rapporti diplomatici e gli accordi bilaterali sono, come già in maniera lungimirante aveva capito il nostro presidente Berlusconi *(Applausi)*, l'unico modo per intervenire in maniera efficace sul controllo dei flussi migratori. Così come non può che farci piacere l'interlocuzione tra lei e la cancelliera Merkel, dato che il problema immigrazione non è solo un problema di accoglienza immediata, ma è una realtà molto più complessa, che necessita l'aiuto di tutti e da tutti i punti di vista. Parlando di diritti sono obbligata a parlare di Turchia. Mi rendo conto che la complessità dei rapporti diplomatici, anche in relazione al piano sull'immigrazione e sui cambiamenti climatici, renda necessaria la ripresa di dialogo e trattative.

Stesso discorso va fatto per la Russia e, di rimando, anche per la Bielorussia. Il disgelo avvenuto tra Putin e Biden non deve far dimenticare all'Europa la propria autonomia rispetto alle decisioni e alle relative sanzioni. Quindi, signor Presidente, credo che questo Consiglio europeo possa essere l'occasione, almeno da parte dell'Italia, per ribadire l'importanza non solo di una comunità economica, ma anche di un'unità di intenti, anche dal punto di vista della tutela e della protezione dei diritti umani e civili. E anche se non è all'ordine del giorno, mi permetta, Presidente, di evidenziare la questione dei diritti delle persone LGBT. A marzo i deputati del Parlamento europeo hanno dichiarato l'Unione europea zona di libertà LGBT, in risposta all'arretramento sui diritti civili in alcuni Paesi, in particolare Polonia e Ungheria. Dunque, signor Presidente, se da un lato siamo tornati a essere forti in Europa, dall'altro le chiedo di far sì che lo diventiamo ancora di più, perché credo fermamente che con lei sia possibile essere un esempio non solo di buona gestione economica e programmatica, ma anche di democrazia e rispetto dei diritti.

Consiglio, come lei ha detto, adesso tocca a noi. Intendo noi come comunità Paese, cioè i cittadini, le Istituzioni, il Parlamento e quant'altro. Non ripeterò - lo sappiamo tutti - che è un'occasione da non perdere. È qui, soprattutto sul piano delle riforme, necessarie come prerequisito, che cominceranno - temo - dei problemi seri. In ogni caso, lei ha toccato i temi che saranno all'ordine del giorno. Le voglio dire tre cose, che tra l'altro stanno nella corposa risoluzione della maggioranza, che sarà depositata tra poco. Migrazioni. A parte qualche accenno, un po' ridondante e molto contorto nelle premesse, relativo alle responsabilità

la persistenza è una virtù. Colgo l'occasione di vedere, come è sempre possibile, la signora Ministro degli interni per dire che forse un elemento di credibilità in più, umano e politico, sta nel fare i compiti a casa nostra. Ora, non so per quale motivo, però delle 207.000 richieste di permesso per lavoro agricolo, come lei ricorda - e sono contenta che ci sia la collega Bellanova,

voglio anche segnalare che è vero che chiediamo alla Turchia più diritti e quant'altro, però non è arrivato il momento di chiedere anche ai nostri colleghi ungheresi e polacchi di essere più coerenti smettendola di usare l'Unione europea come un puro bancomat e violando tutto il resto? Questo, secondo me, è anche un problema di credibilità. Succede che quando incontro...

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentanti del Governo, vorrei rivolgere al presidente Draghi un ringraziamento e poi degli auguri. Il ringraziamento è perché ha contribuito con la sua azione e con questa maggioranza a ridare centralità all'Italia tanto nel contesto europeo quanto nel contesto internazionale più ampio:

sono dovuti alla bellissima promozione a pieni voti che ieri ci ha riconosciuto l'Europa per il Piano Italia domani, che ha avuto un importante successo - ricordiamolo per onestà intellettuale - solo ed esclusivamente grazie a questo Governo. *(Applausi)*. Adesso bisogna andare avanti bisogna farlo secondo due percorsi. Il primo è quello delle riforme, così che si possano accelerare i tempi e migliorare le *performance* di spesa di questi finanziamenti, a cominciare dalla giustizia. proposito, colgo l'occasione per dire che chiunque dovrebbe sostenere i quesiti referendari che la Lega, insieme ai radicali, ha messo su, perché non sono contro qualcuno ma a sostegno di questo Parlamento e di questo Governo. Bisogna riformare la pubblica amministrazione e azzerare il codice degli appalti; occorre inoltre ottimizzare questi investimenti affinché, come ha avuto modo di dire anche lei, presidente Draghi, siano strutturali e non occasionali. Sulle vaccinazioni, la parola data è stata mantenuta: le vaccinazioni vanno avanti così come da programma; bisogna monitorare le varianti e bisogna fare i dovuti complimenti a quell'emblema che oggi è diventato il generale Figliuolo, che gira in lungo e in largo l'Italia, orgoglioso sia della divisa che indossa (che non mette paura ma che rassicura), sia per i risultati importanti che sta portando a casa. Tra le varie cose che ieri ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha anche affermato che l'Italia è stata un esempio di solidarietà. uscendo dalla crisi pandemica, avete ispirato un intero Continente e avete dimostrato qual è il vero significato della solidarietà. Bene, ora noi ci aspettiamo che sia l'Europa

dato un'ulteriore risposta mettendo a disposizione dei Paesi più poveri ben 15 milioni di dosi di vaccini, in modo che tutto il mondo vada avanti più o meno alla stessa maniera. Tornando all'immigrazione, però, l'Europa deve fare presto, perché i numeri sono preoccupanti. Quest'anno,

visto che parliamo di immigrati irregolari o immigrati incontrollati. Vorrei esprimere vicinanza e solidarietà a quel poliziotto che qualche giorno fa, presso la stazione Termini di Roma, ha fatto esclusivamente il suo dovere per tutelare la sicurezza pubblica. *(Applausi)*. Noi ci aspettiamo che quel procedimento penale sia archiviato subito, che vengano indagati altri, ma non chi con onore indossa quella divisa. Nel frattempo, signora Ministro dell'interno, cosa deve fare l'Italia? Non credo debba aspettare l'Europa. Credo che l'Italia debba fare il suo dovere, debba adoperarsi, difendere i suoi confini via terra e via mare, come fanno tanti altri Paesi: la Spagna difende i suoi confini, la Francia difende i suoi confini, Malta difende i suoi confini, la Slovenia difende i suoi confini; tutti difendono i loro confini, non capiamo perché non debba farlo nel frattempo anche l'Italia Il piano Next generation EU parla dell'Italia di domani e noi la intravediamo all'orizzonte, signor presidente Draghi: un'Italia del domani che cammina sulle gambe della fiducia e del coraggio; quella fiducia e quel coraggio che gli italiani hanno dimostrato di avere in questo anno e mezzo difficile. Vediamo un'Italia veloce, efficace, un'Italia giusta, in grado di garantire la coesione sociale, e un'Italia onesta, in grado di investire queste risorse mantenendo fuori tutta la galassia della criminalità organizzata. Questo è il percorso felice e irreversibile verso il quale siamo destinati ad indirizzarci, basta crederci.

Consiglio, ho ascoltato il suo discorso e, a parte complimentarmi per aver dismesso quella politica di adeguatezza e proporzionalità tentennante che non ci avrebbe mai potuto portar fuori dall'emergenza pandemica,

È una sciocchezza in via di fatto prima ancora che di diritto, perché se lei immagina una nave cinese o coreana, che porta 20.000 unità equivalenti si renderà immediatamente conto che non può farsi carico di portare i migranti in Corea, altrimenti è chiaro che quella nave, come tutte le navi in quelle condizioni, tirerà dritto.

risolutezza e determinazione possa cessare il finanziamento alla Guardia costiera libica. Attenzione, il 21 e 22 aprile sono morte 130 persone per l'assoluta incapacità di coordinamento della Guardia costiera libica. Non esiste un coordinamento della Guardia costiera libica e ciò è oggetto di un esposto che anch'io modestissimamente sto contribuendo a firmare e a portare avanti. Come dice infatti anche la Guardia costiera italiana, attraverso il suo rappresentante per le relazioni pubbliche, la Guardia costiera libica non ha

Dobbiamo far tornare in mare la nostra Guardia costiera, al di là delle 12 miglia. Le 12 miglia infatti sono acque territoriali e il soccorso in mare non si fa soltanto nelle acque territoriali, altrimenti, al largo di Ischia, oltre le 12 miglia non dovremmo salvare nessuno.

Queste persone non sono irregolari, sono naufraghi quelli che prendiamo in mare, questa è la più grande mistificazione. Ancora una parola, una sola parola, perché lei, Presidente, ha detto che se le fosse stata posta la domanda, avrebbe risposto.

Mi dispiace, non ho dato a nessuno tempo in più. Può però depositare le sue osservazioni che saranno allegate al Resoconto.

Il MoVimento 5 Stelle continua a ribadire l'importanza di riprendere e rinvigorire il dialogo costruttivo con Mosca affinché si possa consolidare un rapporto proattivo con un attore che resta innegabilmente un *partner* fondamentale per l'Europa sia in termini commerciali che geopolitici. Adottare un approccio di rottura e contrapposizione sarebbe dannoso e controproducente. A fronte dell'oggettivo peggioramento delle relazioni tra Bruxelles e Mosca, su cui ha pesato soprattutto la vicenda dell'oppositore filo-occidentale Navalny, l'Italia, pur senza rinunciare a sostenere sempre il diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani, deve prodigarsi per evitare che il divano tra Unione europea e Russia si approfondisca, mantenendo aperti i canali di cooperazione con Mosca. Per questo attendiamo con trepidazione la discussione della relazione dell'Alto rappresentante e della Commissione sulle opzioni strategiche sui rapporti tra Unione europea e Russia. Presidente Draghi, a mio avviso, l'Italia deve mantenere i suoi tradizionali rapporti di amicizia con Mosca, non solo in virtù dell'interesse economico nazionale e delle intense relazioni commerciali bilaterali, ma anche per la funzione strategica che la Federazione russa svolge nella stabilizzazione di alcune Regioni fondamentali per il nostro Paese. Basti pensare alla Libia, dove il ruolo di Mosca è indispensabile per il buon esito del processo di riconciliazione e pacificazione nazionale. Non possono tuttavia essere ignorate le lacune nella tutela dei diritti umani. Il progressivo restringimento della sfera delle libertà fondamentali in Russia, come altrove, deve destare sempre preoccupazione; diritti e libertà fondamentali che rappresentano i pilastri imprescindibili della cultura dell'Unione europea e del nostro Paese e che, in quanto tali, non sono negoziabili. I diritti umani vanno difesi in quanto valore assoluto e non devono essere strumentalizzati a scopo politico tanto più quando questo può aggravare una situazione già molto preoccupante come quella ucraina, dove rischiamo una nuova guerra alle porte d'Europa con il potenziale coinvolgimento della NATO.

l'opportunità di evitare un eccessivo e rischioso irrigidimento nei rapporti con Mosca. Come ha ricordato nel suo intervento, un ulteriore argomento già ampiamente trattato in precedenza in sede di Consiglio europeo è il rapporto con la Turchia. Nel corso del Consiglio europeo del marzo 2021 era stata accolta favorevolmente la *de-escalation* delle tensioni nel Mediterraneo orientale, ottenuta tramite l'interruzione delle attività illegali di trivellazione e la ripresa dei colloqui bilaterali tra Grecia e Turchia. Come abbiamo più volte sottolineato, il MoVimento 5 Stelle condivide la posizione espressa dall'Unione europea relativamente alla forte convinzione che la Turchia sia un attore essenziale per il mantenimento della stabilità e della sicurezza del Mediterraneo orientale. L'Unione europea e l'Italia hanno un interesse strategico a sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose con Ankara, basate sul dialogo, ma non irreversibili.

ma anche la sistematica repressione del dissenso politico e della libertà di stampa e la persecuzione contro la minoranza curda. Qualora la Turchia consolidasse e mantenesse un atteggiamento positivo, costruttivo e cooperativo, senza intraprendere azioni o assumere posizioni provocatori o lesive del diritto internazionale, essa dovrà essere interlocutore privilegiato sulle questioni della cooperazione nella gestione dei flussi migratori, del contrasto al jihadismo e al terrorismo e dello sfruttamento delle risorse energetiche *off-shore*, evitando di alimentare tensioni con altri Paesi europei. Presidente Draghi, queste sono le criticità che le chiediamo di evidenziare a Bruxelles, al fine di costruire solide basi per l'avvio di una nuova vantaggiosa stagione nelle relazioni euro-turche ed euro-russe. Da ultimo, voglio esprimere la forte preoccupazione del MoVimento 5 Stelle per la gravissima situazione nella regione etiope del Tigray, alla luce del recente *raid* aereo governativo che ha causato la morte di almeno 80 civili. L'Unione europea chieda con forza un immediato cessate il fuoco per fermare questo conflitto, che già sta provocando ondate di profughi. La stabilizzazione dei Paesi di origine dei flussi migratori deve essere una priorità strategica dell'Europa, dal Corno d'Africa al Sahel, dove l'Italia si sta impegnando in prima linea con una delicatissima missione militare antiterrorismo.

Signor Presidente, penso che questo sia davvero un Consiglio europeo di svolta perché viene dopo un G7 in cui gli Stati Uniti sono tornati all'antico. Biden ha rilanciato la via del multilateralismo rispetto all'atteggiamento di Trump, che sarebbe sbagliato definire isolazionista, in quanto era un approccio basato sui rapporti di forza e di tipo *one to one*. Biden ha detto in maniera molto chiara che gli avversari rimangono quelli di prima, intende costruire le proposte e gli approcci con gli alleati storici. Pertanto, rilanciando il metodo multilaterale, lo fa all'interno dell'Organizzazione mondiale della sanità. È bene che le proposte italiane abbiano attecchito e che si vada verso una collaborazione sempre più strutturata e un'attenzione ai Paesi in via di sviluppo, perché questa rimane una delle più formidabili armi diplomatiche per non lasciare campo libero al tentativo di costruire un nuovo ordine internazionale da parte della Cina. Il progetto della Belt and road initiative è legittimo, basta saperlo e comprenderlo. È corretto che la Cina faccia la sua parte. È corretto che Stati Uniti ed Europa reagiscano insieme, con una proposta altrettanto importante e personalmente ritengo che ci si debba concentrare nel dare contenuto alla proposta del Build back better world. Dobbiamo essere capaci, però, di non fare la fotocopia del progetto cinese, dobbiamo invece costruire un progetto complessivo di infrastrutture con le nostre caratteristiche, tipiche dei modelli delle democrazie liberali, spingendo sull'attenzione e sulla tutela dei diritti umani, sul rispetto dell'ambiente e sulla responsabilità sociale delle imprese, altrimenti non si capisce quale sia la differenza. Dobbiamo dimostrare di essere diversi rispetto all'approccio cinese. Il fatto di avere accanto gli Stati Uniti è una buona notizia: con la nostra autonomia, in maniera leale, facendo le nostre battaglie, questo può essere rafforzato e può essere sostenuto, perché si è ritrovata una collaborazione positiva anche grazie al lavoro che avevamo fatto con il precedente Governo e rafforzato da lei e dalla sua credibilità, Presidente. In questa collaborazione fra Germania, Francia e Italia, Turchia, Sahel e Libia, si tengono insieme i rapporti con la Turchia, per i quali noi accettiamo - penso che sia stato questo anche il senso del suo incontro con la presidente Merkel l'altro giorno - di sostenere un investimento importante da parte dell'Unione europea sulla rotta balcanica, con la richiesta di attenzione sulla messa in sicurezza del Sahel, che rischia di diventare la palestra dei fondamentalisti islamici. il traffico d'armi e passa soprattutto il traffico di esseri umani. Quanto alla stabilizzazione della Libia, noi siamo stati i primi ad andare. Lei, Presidente, ha incontrato il suo omologo libico; bisogna muoversi con grande attenzione, con la collaborazione dei Paesi europei. Sull'immigrazione, ha fatto bene a sottolineare che l'ha rimessa al centro dell'agenda politica; è positivo il superamento del Regolamento di Dublino, è positivo il rafforzamento dei corridoi umanitari e dei rimpatri volontari assistiti: noi siamo quelli che li utilizziamo di meno a livello europeo, quindi chiedere maggiori risorse all'Europa per questo modello penso che sia un passo in avanti certamente utile, così come fare accordi di riammissione a livello europeo, perché siamo più forti e più e più credibili. Il punto dolente è certamente quello dei ricollocamenti. Non si va verso la strada dei meccanismi automatici. Penso che a questo proposito dobbiamo dire una cosa molto chiara, Presidente: va riaffermato il vincolo solidaristico, vanno ritrovate le ragioni dello stare insieme, dello stare insieme, di affrontare insieme le grandi sfide internazionali che non siamo più in grado di affrontare, come Stati, da soli. *(Applausi)*. Questo significa dire ai Paesi dell'Europa orientale che se non ci stanno, ci saranno delle sanzioni dal punto di vista delle risorse. La politica di coesione territoriale ha permesso loro di colmare i divari di sviluppo, grazie a noi e grazie alla nostra solidarietà. Adesso è l'ora di dimostrare che anche loro stanno dentro questo vincolo solidaristico. perché se questa non fosse la strada, penso che dovremo - anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa - dire in maniera molto chiara che noi siamo per l'utilizzo delle clausole passerella e per passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata sui temi dell'immigrazione. Penso che questa sia una battaglia che l'Italia Ricordiamoci che l'Unione europea non è solo un mercato unico, in cui le persone e le merci girano liberamente, non è solo uno strumento innovativo e straordinario per affrontare le sfide internazionali che abbiamo davanti e non siamo più in grado di affrontare da ma è anche una comunità di persone che crede in valori e principi che sono alla base della costruzione europea. Ebbene, non possiamo non vedere che in Paesi come la Polonia e l'Ungheria questi principi e questi valori che hanno a che fare con i diritti delle donne, con la libera scelta, con le libertà fondamentali sia messa a rischio. Bene ha fatto ieri il sottosegretario Amendola, non avendo avuto le risposte e i chiarimenti dovuti, a firmare la lettera con gli altri Paesi europei. Questo vale a tutte le latitudini, vale anche nel nostro Paese. Noi abbiamo gli anticorpi necessari, ma non bisogna mai abbassare la guardia e quindi dobbiamo rafforzare anche in Italia gli strumenti - lo stiamo facendo facendo nel Parlamento - per contrastare e lottare contro ogni forma di odio basata sulla discriminazione in base all'orientamento sessuale. Presidente, voglio dire in maniera molto chiara, da parte del Partito Democratico, che auspichiamo, rispetto all'evoluzione in corso, che si guardi a quello che sta facendo il Parlamento, che sarà aperto al confronto, alla discussione, all'ascolto, facendolo nella maniera più corretta possibile, rispettosa delle norme nazionali e internazionali. Vogliamo, con il Governo accanto, ispirarci al principio della laicità: libera Chiesa in libero Stato. Noi ci muoveremo in questa direzione.

Presidente, ho l'onore e la responsabilità di prendere la parola a nome della componente l'Alternativa c'è, che proprio ieri è stata riconosciuta come componente del Gruppo Misto del Senato. Siamo la seconda forza politica di opposizione riconosciuta, composta da 19 parlamentari, l'unica che oggi prenderà la parola per contestare, con spirito critico ma costruttivo, la sua illustrazione di ciò la sua illustrazione di ciò che intende fare nel prossimo Consiglio europeo. Ha parlato, in particolare, di economia e di pandemia. Per questioni di tempo limiterò a questi due aspetti la mia relazione critica. Lei, per quanto riguarda la ripresa economica, ha tracciato un quadro economico che ha definito positivo e di forte miglioramento e crescita. Tuttavia, noi abbiamo una visione molto diversa dalla sua. Siamo fortemente consapevoli che ci sono sei milioni di poveri totali nel Paese e che solo nell'ultimo trimestre ci sono stati 243.000 nuovi disoccupati.

euro all'ora, per chi cerca di difendere i propri diritti del lavoro perdendo la vita e per le famiglie comuni. Ammettiamo per un attimo che il quadro economico, come dice lei, sia veramente positivo. Noi speriamo di sbagliarci ma, se ha ragione lei, allora non dovrebbe avere difficoltà nel riconoscere e rafforzare le tutele del lavoro e, in particolare, non dovrebbe avere difficoltà a posticipare la fine del blocco dei licenziamenti. Vada in Europa e con i suoi omologhi europei trovi modalità per tutelare il diritto al lavoro di tutti coloro che oggi rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Non faccia solo gli interessi di Confindustria, ma anche dei lavoratori e delle classi più deboli. Lei ha

di una politica espansiva europea per i prossimi mesi. Noi non abbiamo bisogno di politiche espansive per i prossimi mesi, ma per i prossimi anni e, almeno, per tutto l'anno prossimo. Quando lei parla di una politica di medio e lungo termine che dovrà tendere alla riduzione del debito, lei dice qualcosa che ci terrorizza. Lei toglie dall'agenda europea il tema della sterilizzazione del debito pandemico. È di questo che deve parlare in Europa; deve andare a dire che tutto il debito che è stato fatto dall'Italia e dagli altri Paesi

prendere la parola oggi - non deve essere considerato e deve essere sterilizzato. Non si deve dire che nel medio e lungo periodo bisognerà ripercorrere quei sentieri di austerità che erano cari ai precedenti Governi. Passiamo al tema della pandemia.

conseguenti alle politiche di chiusura e di vaccinazione. Non menziona mai la questione della stagionalità del virus. questa parzialità e questa mancanza di obiettività nei dati ci preoccupa. Le faccio un caso specifico. Ho chiesto che i dati giornalieri dei nuovi contagi e dei nuovi decessi per Covid siano disaggregati indicando quanti di questi erano stati vaccinati. Questo dato non è presente. Io l'ho chiesto all'Istituto superiore di sanità e al Ministero della salute e non ho avuto risposte. Lei deve dire in Europa che ci siano i mezzi per fornire i dati disaggregati, affinché tutti e la scienza si possa fare un'idea corretta e non funzionale alla narrazione del Governo, come è già avvenuto in passato e come già ci ha fatto vedere purtroppo il capo di Gabinetto del ministro Speranza.

nella parte iniziale della sua relazione, presidente Draghi, lei ha parlato dei rischi che ci sono ancora, pur in un contesto economico positivo:

I mercati hanno già scontato un forte rimbalzo dell'economia nordamericana ed europea, nonché una crescita notevole della domanda globale. I mercati però ora puntano l'attenzione al 2022-2023, cioè alla fine delle politiche straordinarie di stimoli fiscali, di cospicui investimenti di moratorie, dei tassi a zero e di acquisto del debito pubblico, temendo una recessione. Sono timori fondati? Io, presidente Draghi, rispondo che dipende molto da cosa faranno le banche centrali e da come i Governi spenderanno le risorse stanziate a debito. La qualità della spesa, spesa, la qualità degli investimenti, la messa a terra di queste cospicue risorse saranno la chiave di lettura, se abbiamo visto bene e se il nostro ottimismo, che oggi ci vuole, è un ottimismo ben riposto. 191 miliardi e mezzo di debito, con una crescita del PIL, a fine PNRR, cento, non ci pongono nella condizione matematica di poter rimborsare i debiti che abbiamo. Lei lo dice in maniera indiretta nel suo intervento, ma dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. *Gobernar no es asfaltar*, c'è questo famoso brocardo. Chi, come lei oggi, si trova ad avere la responsabilità di governare il nostro Paese, ha anche la capacità di proporre delle soluzioni. È indubbio che c'è una ritrovata fiducia dell'Europa nei confronti dell'Italia. Signor Presidente, senza piaggerie, c'è una fiducia essenziale nella sua persona e di questo dobbiamo essergliene grati. Ci ricordiamo tutti quando, non più tardi di un anno fa, ci rimandarono a casa a fare i compiti, quando rigettarono tutte le nostre proposte senza nemmeno degnarci di considerazione. Signor presidente Draghi,

mandato, Presidente, porti pazienza, lei ha una responsabilità nei confronti dell'Europa: chi governerà l'Europa nei prossimi anni? Presidente Draghi, lei sa che nei Vangeli c'è la parabola dei talenti, per chi ci crede; uno dei peccati gravi che al catechismo ci hanno insegnato è il peccato di omissione. *(Applausi)*. Lei ha una responsabilità Lei ha una responsabilità storica, che ci porta a poter rigiocare, attraverso di lei, un ruolo importante per il nostro Paese; io penso che non le mancherà. Il nostro presidente Berlusconi, sin da subito, dall'appello del Presidente della Repubblica di mettere da parte le logiche di parte e di impegnarci, individuò in lei la figura assolutamente in grado di traghettarci fuori da questa situazione. Toccherà a lei, presidente Draghi, confermare sul campo la fiducia che non solo l'Italia, ma tutta l'Europa le ha confermato. La visita della presidente von der Leyen ieri ne è un'ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno.

approfitto di questa discussione per sottoporre a voi e all'Assemblea due punti di attenzione, uno in una prospettiva di breve e uno in una prospettiva di medio termine. Credo che sia nostro dovere staccarci dalla contingenza e guardare avanti, perché prevenire è certamente meglio che curare, anche se questo - come argomenterò - non significa però che la profilassi possa sostituire o cancellare la terapia e viceversa. Ciò vale sia per il corpo umano, che per il corpo sociale. La riflessione a breve riguarda la strategia di contrasto al Covid-19. A distanza di più di un anno della sua comparsa, possiamo dire di avere a che fare con una malattia estremamente grave e insidiosa, ma che in una grande quantità di casi ha dimostrato di essere curabile, se affrontata per tempo. Ciò non vuol dire ovviamente che non si debba fare tutto quello che si sta facendo, di cui le siamo sinceramente grati, per prevenirla, ma non si capisce perché non si veda un impegno apprezzabile da parte delle istituzioni nel curarla, cioè, per essere inequivocabilmente precisi,

Ripeto, per la massima precisione: mi riferisco alle terapie domiciliari - che dunque non richiedono e in effetti, in moltissimi casi documentati, scongiurano l'ospedalizzazione - e precoci, cioè che non intervengono solo dopo un peggioramento della situazione. Voglio osservare che se nostro Signore, o l'evoluzione naturale - lascio scegliere, perché siamo per la libertà anche di culto - insomma, se qualcuno o qualcosa, ha disposto che il nostro organismo reagisca a certe intrusioni alzando la propria temperatura corporea, un motivo ci sarà e non sarà del tutto sbagliato, visto che da scimmie arboricole siamo diventati individui coscienti. Viene quindi un po' strano pensare che l'unico consiglio che il Ministero, sicuramente popolato da persone coscienti e coscienziose, sta ancora dando a chi ha la sventura di essere attaccato da questa grave malattia, sia quello di aspettare il peggio, reprimendo con antipiretici l'unica reazione naturale del nostro organismo, quando esistono altre strategie terapeutiche sperimentate. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con i pur utili fondi che il PNRR destina al tema della sanità territoriale, tant'è che, anche in assenza di questi fondi, alcuni medici di medicina generale si sono organizzati e reagiscono salvando vite, nel rispetto del giuramento di Ippocrate e nel pieno e legittimo esercizio di un'altra libertà: quella di cura. Anche qui voglio essere estremamente chiaro: non si tratta di promuovere assolutamente il fai da te, come qualcuno ha detto, ma di coinvolgere e valorizzare i medici di base e la loro libertà di proposta terapeutica, basata sulla conoscenza che essi hanno dei loro pazienti. esattamente se non si fa così, cioè se non si promuovono e disciplinano a livello istituzionale le terapie domiciliari precoci, che si incentiva il fai da te, esponendo oggettivamente a rischi. Va però anche detto, *sine ira et studio*, che se va prevenuto il potenziale fai da te dei pazienti, forse andrebbe anche gestito un certo fai da te ministeriale, che ultimamente è parso di vedere ad alcuni nella nota vicenda dei *cocktail*, su cui mi taccio, per carità di patria. Confidiamo in lei perché la razionalità prevalga. Se non dovesse prevalere, temiamo che la strada sia segnata: se non si prevedono nuovi posti letto e non si prevengono le ospedalizzazioni, c'è il rischio che in autunno si debba riprendere la strada delle misure restrittive, nonostante il successo della campagna vaccinale, di cui le riconosciamo il merito. Vengo allo scenario a medio termine, diciamo al 2023, che in qualche modo ci pone in una prospettiva uguale e contraria. Voglio dire che, mentre per il Covid-19 si sta facendo molto per prevenire e meno per curare, nel caso dell'altra infezione europea, l'austerità, si è fatto molto per curare da parte di questo Governo, con due decreti sostegni e altre misure che hanno dato sollievo a cittadini e imprese, come lei ha giustamente rivendicato. Tuttavia, non è forse altrettanto chiaro che cosa si stia facendo per prevenire. Nel 2023 verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale e tornerà, quindi, in vigore il Patto di stabilità, che, come abbiamo capito, non è anche di crescita. Molti, a partire da lei, hanno messo in guardia contro i pericoli del ritorno a uno scenario *business as usual*. Tutti dicono che occorrono nuove regole per prevenire il soffocamento dell'economia italiana ed europea, ma, onestamente, non è ancora del tutto chiaro se ci sia e quale sia la proposta del nostro Governo al tavolo della riforma delle regole. Questa è l'unica riforma veramente indispensabile, senza la quale tutte le altre sono, purtroppo, destinate a fallire, insabbiandosi nella stagnazione economica. Nessuna riforma delle regole sarà credibile né efficace se non abbandonerà il riferimento al PIL potenziale e all'*output gap*, la cui distorsione prociclica è ormai comprovata da una ampia letteratura. La prevenzione, in questo e in altri casi, passa da qui: dall'abbandonare definitivamente regole assurde, come il *calendar provisioning*, i cui gravissimi limiti abbiamo denunciato per primi, inascoltati. Confidiamo che lei ci stia lavorando. In sintesi, un maggior equilibrio tra profilassi e terapia ci aiuterebbe in entrambi i casi. Confidiamo in lei perché questo maggior equilibrio possa prevalere, qui e a Bruxelles. Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Presidente del Consiglio, tra i temi da lei trattati oggi c'è la ripresa economica. Lei domani sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo ed è davvero un bel momento per arrivarci, dopo l'approvazione del PNRR italiano da parte della Commissione europea, il cui importo, che ammonta ad oltre 200 miliardi, rappresenta più di un quarto di tutti i fondi che l'Europa ha messo a disposizione del Next generation EU (o *recovery fund* che dir si voglia). È innegabile che questa approvazione segni un grande riconoscimento per il lavoro fatto dal nostro Paese e costituisca l'ennesima conferma che il percorso indicato all'Europa dal presidente Conte per affrontare la crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia fosse il percorso giusto, lungimirante e innovatore, anzi rivoluzionario. Ora sembra tutto facile, tutto scontato, tutto quasi elementare, ma poco più di un anno fa, nel pieno della pandemia, non lo era affatto. C'era uno scontro politico duro tra i Paesi cosiddetti frugali, i rigoristi, i sostenitori dell'*austerity* da una parte e chi, dall'altra parte, guardava lontano e voleva un'Europa diversa, più giusta, più solidale, più inclusiva. Noi del MoVimento 5 Stelle ci battevamo per un'Europa nuova che mettesse le persone al centro dell'azione politica. Ambivamo a una vera Unione di Paesi moderni e democratici, che volessero stare insieme per fare sviluppo sostenibile e per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Oggi come allora non volevamo un'Europa come coacervo di interessi di affaristi e di banchieri. Ricordo agli smemorati che nei momenti più drammatici dall'inizio della pandemia

In quei momenti, alcuni politici olandesi, amici e alleati di Salvini e della Meloni, urlavano: non un centesimo all'Italia. Ora fa quasi sorridere. Sembra passato un secolo e, invece, è passato solo un anno e questi progressi giganteschi li dobbiamo al presidente Giuseppe Conte e al suo Governo. L'approvazione del PNRR, il cui testo è pressoché identico, secondo alcuni al 95 per cento, a quello predisposto dal precedente Governo, è il riconoscimento definitivo del grande lavoro fatto dal Governo Conte II, di cui giustamente quello attuale segue le orme. Grazie a questo enorme lavoro, a luglio arriveranno in Italia 25 miliardi. Ossia la prima *tranche* del *recovery fund*. Quindi, chi per mesi ha urlato falsamente che eravamo in ritardo, spero chieda scusa o taccia per un po'. Se tutto questo lo dicessi solo io o lo dicesse soltanto il MoVimento 5 Stelle, potrebbe essere scambiato per una visione di parte. Invece lo ha affermato, alcuni giorni fa,

Credo che sia necessario ricordare tutto questo perché in quest'Aula, ma anche in alcune Commissioni permanenti, qualcuno ha voluto sminuire l'enorme lavoro fatto negli scorsi mesi, parlando di una formuletta: secondo un senatore di Fratelli d'Italia gli oltre 200 miliardi del Next generation EU sono arrivati in Italia grazie a una formuletta. So che è assurdo, ma è stato affermato qui, in Commissione bilancio, l'ho sentito con le mie orecchie. Vorrei porre allora dei quesiti agli esponenti del centrodestra. Se era così facile, perché tutto ciò non è stato fatto nel 2008-2009, quando l'Europa fu colpita dalla crisi dei mutui *subprime*? Perché non è stato fatto nel 2011 (Governo Berlusconi), quando l'Italia, in piena crisi sul debito sovrano, era attaccata dalla speculazione internazionale? centrodestra, applicare la cosiddetta formuletta, perché, invece di ottenere - come oggi noi siamo riusciti - 230 miliardi, di cui 80 a fondo perduto, i Governi dell'epoca si sono piegati all'austerità imposta dall'Europa, che ha creato oltre 5 milioni di poveri in Italia, che ha fatto morire centinaia di migliaia di aziende, che ha tagliato le pensioni di milioni di italiani, che ha impoverito un'intera Nazione, che ha precarizzato milioni di giovani?

dai Presidenti uscente ed entrante della BCE, in cui si elencavano le riforme lacrime e sangue che l'Italia avrebbe dovuto applicare e poi in effetti ha applicato? Avete quindi impoverito il Paese, avete distrutto la vita di milioni di italiani, salvo poi dare la colpa al senatore Monti da voi stessi sostenuto. Concludo dicendo che ora siamo in una fase nuova grazie alle battaglie del MoVimento 5 Stelle e alla nostra forza parlamentare. Confidiamo che le nostre proposte politiche diano frutti ancora più ricchi. fiduciosi che vengano messi in discussione e cambiati per sempre alcuni baluardi di quell'epoca, quali il pareggio di bilancio in Costituzione, il meccanismo di stabilità, gli assurdi e non scientifici parametri sul debito e sul *deficit*. Siamo convinti che una nuova Europa sia alle porte, l'Europa dello sviluppo, della solidarietà, della giustizia sociale, dei cittadini e degli Stati, non certo l'Europa dei banchieri e delle *lobby*. Confidiamo di fare questo tutti insieme. Signor Presidente, signor presidente Draghi, esponenti del Governo, onorevoli colleghi, siamo convinti di una cosa: bisogna intervenire su quei fattori che provocano le migrazioni. È necessario combattere le cause dei processi migratori e non i migranti. Bisogna combattere allora guerre, carestie, stravolgimenti climatici, povertà, quei fattori che inducono centinaia di migliaia di persone a mettersi in fuga in cerca di prospettive più promettenti. Bisogna investire nei luoghi di origine, cosicché le persone trovino opportunità di lavoro nelle loro terre e non siano costrette ad andarsene. Draghi, la sua proposta al Consiglio europeo di affrontare tutti insieme alla radice la questione migratoria, come fosse una questione di politica estera per l'Europa e non solo di politica interna, può essere strategica, perché ci consente di spostare il baricentro e di puntare l'attenzione sui Paesi di partenza, nel tentativo di creare lì le condizioni per cui si possa smettere di emigrare in massa e si possano evitare le troppe stragi nel Mediterraneo. Insistiamo, cioè, sulla necessità di intervenire a monte, così da non limitarci a piangere i morti in mare, investendo in via anticipata per creare sviluppo e ridurre le partenze. È quindi un vero e proprio cambio di paradigma, che non può però di certo diventare una scusa per alcuni Paesi per sottrarsi ai propri obblighi nell'accoglienza dei profughi già arrivati. Ecco che a Bruxelles bisogna continuare a pretendere una gestione condivisa, attraverso una riforma del Regolamento di Dublino, che li ripartisca in modo equo tra i diversi Stati, imponendo a coloro che si rifiutano di accogliere i migranti di farsi almeno carico dei costi per la difesa delle frontiere esterne. Girarsi dall'altra parte di fronte alla sfida migratoria e lasciare da soli i Paesi di frontiera è un atteggiamento che non può essere tollerato ulteriormente. Paesi come l'Ungheria, che da tempo snobbano il *dossier* migrazione, devono essere costretti a cambiare atteggiamento. È giusto insistere su una strategia europea di ingresso legale nei nostri Paesi e di sostegno ai rimpatri volontari, favoriti anche da adeguati incentivi, erogati alla luce di intese e di partenariati stilati *ad hoc* con vari Paesi, a partire dalla Libia e dalla Tunisia, dal Sahel e dal Corno d'Africa. Insomma, un cambio di visione che impegni tutti i Paesi europei ad affrontare il problema sin dalle sue fondamenta; una visione, dunque, che può segnare una svolta importante nel far fronte al fenomeno migratorio, rimettendo lo sviluppo del continente africano all'ordine del giorno dell'agenda europea, esattamente come l'Italia aveva già cominciato a fare con i Governi Renzi e Gentiloni Silveri. Adesso serve un'azione coordinata da parte di tutta l'Unione europea, così che possa avere un impatto significativo; perché è una questione di umanità, ma anche di buon senso. Entro la fine di questo secolo, il continente africano vedrà quadruplicare i propri cittadini, il che significa che esprimerà il 40 per cento dell'intera popolazione mondiale, tra l'altro con un'età media molto giovane, attorno ai vent'anni, rispetto invece a una diminuzione della popolazione in Europa, sempre più anziana. Ecco perché serve un nuovo approccio rispetto alle politiche migratorie. È positivo che sia l'Italia a rendersene artefice, perché il futuro di un continente come l'Africa non può essere l'emigrazione, soprattutto un'emigrazione selvaggia e pericolosa, con la quale ogni giorno nel Mediterraneo sono in pericolo migliaia di vite umane. Bisogna creare nella stessa Africa sufficienti possibilità di crescita, così che ne traggano beneficio le persone sul posto, ma anche coloro che avranno avuto la capacità e l'intelligenza di investire in quel continente, Europa in testa. Ecco che un cambio di approccio, che declini la politica migratoria come politica estera, senza per questo tralasciare le battaglie storiche in materia, può essere una strategia utile per fare passi avanti su più fronti. Anche perché lo scacchiere internazionale si sta ridefinendo. Assistiamo ad atteggiamenti sempre più aggressivi, anche alle soglie di casa nostra, da parte di Paesi come la Turchia, la Russia, la Cina, che sempre più frequentemente calpestano diritti e libertà interne, ledono gli interessi di altri Stati attraverso attacchi illeciti e vengono meno al rispetto del diritto internazionale. L'Unione europea non ha interesse ad accettare tutto questo; anzi, a partire dal Mediterraneo, è necessario favorire processi di stabilizzazione a livello internazionale. Ecco che è opportuno che l'Europa continui ad arrivare a una netta condanna delle violazioni dei diritti, siano essi civili o internazionali, e inviti ad astenersi da azioni unilaterali provocatorie nei confronti di altri Stati. Insomma, signor Presidente, siamo alla vigilia di un Consiglio europeo importante, che coincide con il battesimo del Next generation EU, la più brillante risposta che l'Europa potesse dare a una drammatica pandemia come quella da Covid-19, che ha rischiato di mettere in ginocchio il mondo intero. La visita ieri a Roma della presidente von der Leyen ha sancito anche per il nostro Paese il fischio di inizio di una nuova straordinaria partita, una ricca stagione di investimenti dedicati alla ripresa e alla realizzazione di quelle riforme di cui il Paese ha bisogno da decenni. È una scommessa e noi siamo contenti, signor presidente Draghi, che sia lei, a nome dell'Italia, a giocare questa partita in Europa. Buon lavoro e grazie. Signor Presidente, signor presidente Draghi, il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno reca proprio l'aggiornamento delle valutazioni concernenti la situazione epidemiologica e vaccinale e gli sforzi di coordinamento in risposta alla pandemia da Covid-19. Lei, Presidente, secondo

è un po' diverso da quello che probabilmente le viene relazionato. Noi abbiamo una squadra di governo della pandemia che, rispetto a quello che è accaduto dai primi mesi del 2020, ha collezionato una serie di dati negativi e *record* negativi, un *palmarès* di difetti che avrebbe suggerito

alla storia: la necessità di testare la presenza del virus nella popolazione (il *testing*); la necessità di tracciare i positivi in modo da isolare i focolai; la necessità di trattare il virus con adeguate terapie, prime fra tutte quelle domiciliari. Ebbene, signor Presidente, rispetto a tali macrocolonne per affrontare la pandemia, la nostra Nazione ha fallito miseramente su tutte e tre.

Rezza si è svegliato come Biancaneve dopo un lungo letargo e ha detto che l'errore

Quindi, la parte che riguardava la ricerca del virus nei non sintomatici è ancora oggi fallita e non la stiamo facendo. Signor Presidente,

Chi deve venire a fare il sequenziamento dei nostri positivi e dei nostri ipotetici focolai di varianti? È questo il vero grande pericolo rispetto alla vaccinazione di massa che stiamo facendo.

Ci è stato raccontato che, a causa dei grandi numeri che hanno superato ampiamente le dimensioni previste del fenomeno, il tracciamento si è perso. Se è perso. Se si è perso il tracciamento con i grandi numeri, oggi che i numeri sono assolutamente inferiori riprendiamo quel tracciamento o pretendiamo di rifare il tracciamento con la *app* di Conte e di Arcuri? Lo dico al collega che è intervenuto poco fa: abbiamo visto tranquillamente quello che è accaduto. Rifacciamo un altro strumento di tracciamento? E soprattutto, aumentiamo le strutture di farmaco-vigilanza e di vaccino-vigilanza per avere contezza e analisi precise degli eventi avversi? Gli eventi avversi ci sono e vanno valutati, tracciati e affrontati. terzo problema è quello che ha perfettamente illustrato il collega Bagnai nel suo intervento, ossia quello del trattamento. Il vaccino, infatti, non è il trattamento della pandemia ma la profilassi

Ormai la comunità scientifica ci dice unanimemente - se vuole le fornisco i dati, ma li chieda al qui presente collega Sileri, che ne è assolutamente al corrente - che il vaccino a RNA messaggero non copre dalla possibilità di infettare.

e una inutile cura certa. Inoltre, signor Presidente del Consiglio, dal punto di vista etico io un problema me lo farei, perché vaccinare i minori per proteggere gli adulti

sono tre anni in più rispetto al 1995; la percentuale di nati da genitori coniugati è del 33,4 per cento, era

L'Italia è legata all'Europa in maniera indissolubile in questo momento. Devo dire che il viaggio di cui eri la Presidente ha parlato è iniziato un anno e mezzo fa ormai. È iniziato da quando si è deciso di condividere con tutti gli Stati membri i passaggi per contrastare l'epidemia,

Certo che ce la dobbiamo meritare e allora è bene strutturare l'economia, così come è stato fatto, ma questo stesso proposito deve essere anche mantenuto per la sanità. di un tema fondamentale. La boccata di ossigeno del Piano apre infatti una stagione di investimenti mai avuti e mai visti in sanità, sui quali noi, come Parlamento, saremo vigili per vedere effettivamente il loro utilizzo. Come ha detto anche lei, controlliamo tutto ciò che avverrà. Benissimo, dobbiamo però già adesso pensare di trovare risorse per evitare di essere sempre in emergenza perché dobbiamo ovviamente trovare e stabilizzare il personale sanitario che noi abbiamo previsto nel PNRR e che al 2026 abbiamo bisogno di mantenere in essere; pensare già a superare i tetti di spesa, che sono stati una tenaglia importantissima, che ha smembrato tutti i nostri servizi e il Sistema sanitario nazionale, credendo già nelle prossime assunzioni, oltre ad una buona programmazione delle figure professionali di cui noi avremo bisogno e che saranno necessarie per non trovarci impreparati.

Misto. Siamo confortati peraltro dal fatto che rispetto a pochi mesi fa, quando abbiamo iniziato ad agire politicamente, sono quasi tutti diventati europeisti e quindi forse abbiamo seminato bene, forse qualcuno è rimasto convinto delle argomentazioni che abbiamo sempre posto davanti alla nostra azione politica e cioè che il campo da gioco per l'Italia è quello europeo e non vale la pena di sprecare tempo e forze in campi secondari e provinciali. Abbiamo quindi tempo per approfondire i temi economici; prendiamo come auspicio le sue rassicurazioni sul rialzo dell'inflazione *core* nelle macro aree europee e americane, come un rischio non impattante sulla sostenibilità del debito pubblico italiano, continua a crescere, così come sul Patto di stabilità e crescita che, perlomeno fino al 2023, nella forma precedente non precedente non sarà rimesso. Mi concentro sul tema delle emigrazioni nella duplice veste di immigrazioni ed emigrazioni. Le immigrazioni

importante, non possa limitarsi a mettere dei soldi sul tavolo, ma debba offrire qualcosa di più. Alla sponda Sud del Mediterraneo

dell'European forum sulla possibilità di dirigere la svolta *green* anche in questi Paesi. Dobbiamo poter offrire sviluppo culturale e democratico, senza naturalmente rinnegare i nostri valori principali.

Tuttavia, si può ancora fare meglio. Per quanto riguarda la dimensione interna, abbiamo letto il *draft* del comunicato finale del Consiglio europeo. Non riteniamo sufficiente il rinvio all'autunno 2021 della presentazione, richiesta alla Commissione europea, da parte del Consiglio di piani di azione per la gestione. Capiamo benissimo le condizionalità

(Francia, Malta, Cipro e Grecia), l'impegno del Governo italiano dovrebbe essere nel senso di ottenere qualche cosa prima dell'autunno. dell'autunno. C'è tra l'altro la possibilità di utilizzare la Conferenza sul futuro dell'Europa, che è partita adesso e di cui noi europeisti siamo stati i primi a parlare in Italia il 10 marzo, quando sono stati firmati a Bruxelles i trattati istitutivi, per inserire il principio dell'eventuale modifica dei trattati. A noi interessa modificare il Trattato di Dublino e dobbiamo essere audaci. Presidente Draghi, alla Camera lei ha detto: chi avrebbe pensato, qualche mese fa, che si sarebbe arrivati al debito comune. Noi possiamo essere così audaci da pensare che la Conferenza sul futuro dell'Europa sia un esercizio utile per arrivare alle modifiche dei trattati. Da ultimo, mi soffermo sul tema dell'emigrazione italiana. Grazie per aver accennato all'importante comunità italiana in Germania e Spagna nei suoi viaggi. L'Unione europea dovrà negoziare nuovi accordi

presidente Draghi, la ringrazio anzitutto per la sua relazione, che ho apprezzato e condiviso punto per punto. La pandemia che ha sconvolto il mondo ci impone tutt'ora di inserire come punto fondamentale nell'agenda politica la lotta al virus. Sarà quindi imprescindibile nel prossimo Consiglio europeo ribadire l'importanza e la necessità, anche per i prossimi mesi, di un coordinamento a livello europeo nel contrasto al Covid-19. La solidarietà internazionale per migliorare l'accesso ai vaccini dei Paesi rimasti indietro sarà l'unico modo per fermare il virus e garantire a tutti la sicurezza in materia sanitaria. La comunità scientifica ci ha più volte spiegato come più esso si diffonde, più si generano varianti. L'Europa quindi deve muoversi nel segno del pragmatismo, tenendo conto inoltre che Paesi come Russia e Cina stanno di fatto utilizzando i vaccini come arma geopolitica. Mi permetta poi una riflessione in continuità con quanto emerso durante il G7 sul ruolo della Cina. Sarà complicato accertare la sua responsabilità nella pandemia *(Applausi)*, ma con sicurezza sappiamo che la Repubblica popolare cinese è colpevole di avere nascosto per mesi la verità sul virus. Sappiamo che non rispetta i diritti dei lavoratori, che rinchiude nei *lager* gli oppositori, che perseguita le minoranze. Quindi, Presidente, anche se al prossimo Consiglio non si discuterà in modo puntuale della questione Cina, le anticipo che riteniamo necessario frenare sull'accordo tra Europa e Cina sugli investimenti; un accordo poco chiaro e definito, poco conveniente per il nostro Paese e che suscita diverse perplessità. Allo stesso tempo, in seguito all'incontro tra Putin e Biden, pensiamo sia importante riprendere un dialogo strategico Europa-Russia, non solo perché le sanzioni hanno danneggiato il nostro tessuto economico, ma anche ai fini della lotta al terrorismo e perché interfacciarsi con la Russia significa impedire che l'abbraccio tra Mosca e Pechino diventi definitivo. Per quanto riguarda l'Africa, è fin troppo chiara l'importanza di un intervento più incisivo dell'Europa nel Mediterraneo; il fenomeno delle migrazioni di massa interessa da troppi anni il nostro Paese senza che l'Europa abbia fatto significativi passi in avanti. Presidente, la sua è una voce autorevole in Europa. Combatta affinché i Paesi membri comprendano che Lampedusa non è solo terra di confine italiano, ma confine d'Europa. La redistribuzione dei migranti è un atto di giustizia dovuto, a cui i Paesi europei non possono ancora sottrarsi. Al contempo, occorre che l'Europa si occupi davvero di Africa. La parola «cooperazione» è la chiave. Sono passati troppi anni da quel lontano 2011, in cui la Libia è stata attaccata militarmente con le conseguenze che paghiamo ancora oggi. All'epoca, il presidente Berlusconi aveva capito come solo con accordi di partenariato stabili e reciprocamente vantaggiosi si sarebbe potuto dare un sostegno alle economie dei Paesi africani e l'accordo con la Libia ne fu un chiaro esempio. Non possiamo, quindi, che essere soddisfatti del nuovo approccio del Governo, che per questa via più complicata, ma senz'altro più feconda - sta provando a ricucire solidi rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il controllo del flusso delle partenze dei migranti sarà realmente possibile solo assicurando sviluppo ai Paesi di partenza. Se la Germania guarda alle sue rotte e all'accordo con la Turchia che in questi anni ha pesato ben sei miliardi sulle casse comunitarie, noi dobbiamo guardare verso il Mediterraneo e agli accordi con Libia e Tunisia. A questo riguardo, Presidente, nella risoluzione che voteremo più tardi ho chiesto al sottosegretario Amendola, che ringrazio per l'eccellente lavoro svolto, di inserire un passaggio a cui tengo particolarmente. In questa c'è scritto che occorre assicurare che nei partenariati strategici dell'Unione europea con i Paesi dell'Africa del Nord siano garantite adeguate misure di sicurezza alle imprese che operano nel Mediterraneo. Solo pochi mesi fa, infatti, alcuni nostri pescatori sono stati sequestrati dai libici e non è stato un caso isolato (chiedo al Presidente del Consiglio e anche alla ministra Lamorgese di ascoltarmi).

mettere a rischio la loro stessa vita. Mi auguro che anche lei, Presidente, possa prendere a cuore questo punto e lo sottoponga ai *partner* europei. È giusto, inoltre, porre il tema del rispetto dei diritti nei confronti della Turchia, certo, ma anche e soprattutto nei confronti dei Paesi dell'Europa. Per questo esprimo forte preoccupazione per la nuova legislazione ungherese contro la comunità LGBT: se Ungheria o Polonia non si fanno scrupolo a ricevere i fondi europei, dovrebbero allo stesso modo rispettare i valori e i principi europei. Da ultimo, le nostre imprese, i cittadini, le famiglie sono ancora provati dalla crisi e occorre assicurare loro risorse finanziarie che forniscano dovute risposte anche nei prossimi mesi. La pandemia ha posto l'Unione davanti a una scelta: se essere solo mera burocrazia o compiere ulteriori passi in avanti per diventare una grande e forte realtà. Il Patto di stabilità è sospeso fino al 2022. Impegniamoci affinché nel 2023 i vecchi parametri, figli di altri tempi, siano rivisti, cancellando l'Europa dell'*austerity* per proseguire sulla via dello sviluppo e della crescita.

Signor Presidente, presidente Draghi, facevo una riflessione poco fa ascoltando le parole di chi mi ha preceduto e, in particolar modo, quelle del professor Bagnai. Questa è una stagione nella quale dobbiamo avere necessariamente lo sguardo teso al futuro pensando bene che ciò che stiamo facendo ovviamente avrà un riverbero ben oltre questa generazione e si proietterà sulla prossima. Le riforme, che sono ovviamente parte fondante rispetto alla sua azione di Governo e alle quali ovviamente abbiamo aderito proprio per la necessità di dare slancio al nostro Paese,

sfugge totalmente a una revisione o a una considerazione da parte di Bruxelles di quanto sarebbe necessario riformare la stessa Unione europea. Ci sono regole di base che è evidente che facevano fatica a funzionare prima ci sono regole di base che è evidente non ci possono garantire stabilità in futuro. E, vivaddio, lo diciamo anche in questa circostanza: l'Unione europea, come qualsiasi Stato, non può essere la sommatoria di tanti interessi particolari, ma deve necessariamente crescere e diventare finalmente qualcosa che ha utilità generale; altrimenti, tutto ciò non ha senso e si è semplicemente una proiezione di un interesse nazionale, magari, nel caso specifico di quello tedesco. tedesco. Su queste cose una riflessione va fatta in termini di democrazia e anche in termini delle stesse istituzioni che rappresentano i cittadini. Noi, infatti, oggi abbiamo un'Unione europea nella quale i cittadini sono rappresentati esclusivamente nel Parlamento, che peraltro è marginale o non principale rispetto alla stessa azione di fare norma. Su queste cose una riflessione la deve portare. È riuscito a imporre all'agenda europea il dibattito sui migranti. Ne siamo soddisfatti, ma occorre anche che l'Unione europea si impegni a un dibattito serio, compiuto, completo e non marginale rispetto all'autoriforma della stessa; altrimenti, tutto ciò di cui parliamo oggi rischia di scontrarsi poi con le frustrazioni che si proiettano sulla nostra popolazione. Presidente, dobbiamo anche ricordarci che in questo momento dobbiamo confrontarci con situazioni ben più ampie, anche rispetto all'Unione europea. Penso ai rapporti economici con la Cina, l'unico Paese che nel corso della pandemia non solo ha tenuto il proprio bilancio in attivo, ma ha accresciuto ancora la propria capacità di penetrazione. Ciò non può essere fatto che attraverso una seria politica economica e, quando serve, di protezione rispetto a penetrazioni che troppo spesso e volentieri sono state descritte come un'opportunità per l'Italia. attenzione. Ha detto prima che in questo momento domande e offerta mettono in difficoltà le nostre strutture produttive, fino ad arrivare anche al rischio di un'impennata inflazionistica. corretto ciò che lei dice e, cioè, che va gestita e tenuta sotto controllo; altrimenti, la stessa carenza delle materie prime che abbiamo voluto richiamata nella proposta di risoluzione e che troppo poco finora è stata oggetto di dibattito in quest'Aula ci creerà dei problemi enormi perché la competitività del nostro Paese non è solo in funzione delle regole che diamo, ma anche dei costi cui le nostre imprese sono sottoposte.

«Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli». Queste parole pronunciate da lei qualche tempo fa sono state da noi particolarmente apprezzate, anche perché hanno tracciato una linea netta sull'obiettivo di Governo. Occorre impegnarsi anche a livello europeo affinché ci sia una revisione delle singole normative fiscali e affinché quel *dumping* che ancora esiste all'interno dell'Unione europea non continui a mettere il nostro Paese in una situazione paradossale in cui le imprese italiane più grandi, grandi, che non hanno vincoli a restare e vanno dove vogliono, smobilitano e spostano la loro sede fiscale o amministrativa in Stati sempre all'interno dell'Unione europea dove la fiscalità - sappiamo - essere molto più vantaggiosa rispetto a quella italiana. Presidente, parallelamente occorre una riforma fiscale in Italia. Su questo Su questo non abbiamo alcun dubbio. Occorre in questo momento dare agli italiani la certezza che fare impresa non è un lusso; fare impresa non è un ostacolo, ma una necessità. Spendere i soldi per creare crescita e occupazione è certezza che in futuro saremo in grado di ripristinare quel debito e di restituirlo. Su questo ovviamente anche all'interno del dibattito europeo la sua voce sarà sicuramente forte. Vede, Presidente, nella proposta di risoluzione che ci apprestiamo a votare fra poco abbiamo voluto che al tema immigrazione fosse inserita una specifica nota: pertanto fondamentale, nelle more di una riforma organica delle politiche di contenimento dell'immigrazione e del superamento di Dublino, assicurarsi che gli Stati di bandiera delle navi europee che effettuano operazioni di salvataggio in mare, collaborino all'individuazione di un porto di sbarco e si assumano la responsabilità dell'accoglienza delle persone soccorse». Il tutto «nel rispetto delle convenzioni internazionali sul diritto del mare». È un'assunzione di responsabilità alla quale dobbiamo chiamare tutti gli altri Paesi europei, perché deve finire quel meccanismo che ha visto navi battenti bandiera di altri Paesi europei fare l'ultimo miglio degli scafisti e poi scaricare, come fossero merce, i migranti in Italia. Noi siamo al Governo per impedire che tutto questo avvenga e sappiamo che...

Signor Presidente, signor presidente del Consiglio Draghi, colleghi, membri del Governo, siamo nuovamente - perché questo è un appuntamento periodico - in procinto di un un incontro europeo, uno di quelli importanti. Abbiamo già ottenuto dei buoni risultati, ma domani si riprenderà a parlare di temi forti, come la ripresa economica e tutta la gestione della fase post-pandemica, anche se la pandemia ancora non è proprio sconfitta. Si parlerà anche di relazioni internazionali: i temi sono quelli legati alla Turchia e alla Russia. Ultima, ma non ultima (almeno dal mio punto di vista), finalmente si ritorna a parlare della questione migrazioni e asilo. È dal 2018 che in un Consiglio europeo non si trattava questo importante tema, che vede la nostra Nazione come una delle più "impattate" da questa problematica. del Consiglio, mi permetto di uscire un attimo fuori dal tema e, prima di affrontare l'argomento migrazioni, di provare a fare delle sollecitazioni. Oltre alla tematica legata al MES, spesso veniva utilizzato il tema dello *spread* come maglio per attaccare i precedenti Governi. Mi permetto di ricordare a lei, ma anche ai colleghi, che, quando è iniziata questa legislatura con il Governo Conte I, abbiamo trovato uno *spread* a oltre 230 punti base; dopo il Conte I e il Conte II glielo abbiamo consegnato a circa 130, perciò l'abbiamo fatto scendere di oltre 100 punti. da 130 siamo a circa 105 nella chiusura odierna; però non si parla più di *spread* e non si usa più lo *spread* come maglio per attaccare il Governo. Io ora le chiedo e mi aspetto - lo dico sinceramente - che con la sua attenta guida questo *spread* si possa avvicinare allo zero. Perciò le chiedo di fare un passaggio anche su questa tematica, sebbene non strettamente legata all'incontro del prossimo Consiglio europeo. Un altro tema, che è stato messo in luce anche dalla collega Masini e sul quale le chiedo magari di fare un breve passaggio, è quello legato alla normativa sull'omotransfobia; un altro tema a noi caro e alla ribalta non solo a livello nazionale, ma anche a livello di Unione europea. Lei sa benissimo che alcuni Stati, che sono in contrapposizione o contrari alla linea nazionale sul tema migrazione, hanno una posizione molto critica (non voglio usare termini decisamente più calzanti e forse più appropriati); questa gente evidentemente ha un approccio democratico diverso dal nostro. Il rispetto dei diritti delle persone deve essere sempre messo al centro e non usato per beghe politiche.

Sentiamo giornalmente che Lampedusa, Porto Empedocle, Pantelleria e tanti dei nostri porti di primo approdo vengono "impattati" da migliaia di

mi dispiace dire - ma la voglio informare di questo, signor Presidente - che coloro che gestiranno la presidenza di turno dal primo luglio, cioè gli sloveni, hanno già manifestato in maniera chiara la loro posizione, perfettamente in linea con i cosiddetti Paesi di Visegrád. Perciò, mi dispiace dirlo, ritengo che anche per il prossimo semestre, sul tema dell'immigrazione, si continuerà a prendere tempo, così come hanno fatto, in precedenza, anche altri due Stati. Signor Presidente, in quell'occasione mi hanno dato soltanto un minuto e mezzo per esprimere la posizione italiana, ma in quei consessi internazionali

vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere generale, prima di rispondere, spero puntualmente, ai vari interventi. Prima di tutto ringrazio tutti voi per le espressioni di stima e di incoraggiamento: sapere che c'è il sostegno di gran parte di questa Camera è la maggiore fonte di forza, per chi deve andare fuori, ma anche per chi deve stare qui e affrontare un programma difficile e urgente.

che l'atmosfera generale è cambiata. È cambiata per moltissime ragioni. La prima è che le economie vanno bene: in alcuni casi benissimo, in altri bene. ragione è che c'è sollievo, perché l'epidemia sembra essere meno grave, sembra essersi attenuata. Il terzo motivo di sollievo è il passaggio da Trump a Biden. Il quarto motivo, in un certo senso conseguenza del terzo, è che è ripresa l'opera di ricostruzione di quell'edificio basato sul multilateralismo, sull'equità, sui negoziati, sui compromessi, sui quali sono stati creati lo sviluppo e la prosperità dal secondo Dopoguerra. Questa è l'atmosfera generale in cui stanno avvenendo oggi le discussioni. terza constatazione, che un po' ho fatto anche stamattina alla Camera, è che, ascoltando tutti i vostri interventi, appare che oggi siamo tutti europei. Se si confronta l'atmosfera di oggi nei confronti dell'Europa con quella di circa sei mesi fa, per non parlare di un anno fa, prima della presentazione del PNRR da parte della Commissione, si vede l'enorme differenza. Ma perché? Questo senso di una maggiore appartenenza all'Europa da parte nostra trova, in un certo senso, rispondenza nel fatto che anche i Paesi membri oggi si rendono conto che, per affrontare sfide di questa dimensione, non si può stare da soli. Bisogna farlo insieme. Infatti, appena chiesto di mettere all'ordine del giorno il tema migrazione, che, come dicevo prima, è dal giugno del 2018 che non veniva più messo all'ordine del

Quindi, in un certo senso, i vostri interventi di oggi e l'atteggiamento generale dei membri del Consiglio europeo marciano di comune accordo verso un maggiore e più forte riconoscimento dell'Europa come entità di riferimento.

non è esattamente vero che tutti i problemi stanno ancora lì. Tanto è stato fatto. È stato fatto un decreto semplificazioni, è stata fatta una riforma della pubblica amministrazione, è stata fatta una riforma del reclutamento nella pubblica amministrazione. Vi sarà presto una legge sulla concorrenza. Sulla riforma della giustizia, lei ha giustamente richiamato la necessità che sia fondamentale, che sia profonda e che non sia, come ha detto, un pannicello caldo: vedremo. Prima della fine del mese sarà presentato il disegno di legge delega sulla riforma del codice degli appalti e delle concessioni.

secondo luogo, non è che in Libia non abbiamo carte da giocare. Ne abbiamo e, secondo me, ne abbiamo almeno quanto tutti gli altri attori, che devono e vogliono essere coinvolti in quella parte del mondo. L'attore che avrebbe più carte da giocare non vuole essere coinvolto in quella parte del mondo: questo è stato anche oggetto dei colloqui avuti in Cornovaglia. Quello che però si sta cercando di fare è sollecitare l'azione dell'Unione europea come tale sotto l'auspicio delle Nazioni Unite e a quel punto vedere se gli Stati Uniti possono affiancare o comunque essere favorevoli all'azione delle Nazioni Unite in quella parte del mondo, di nuovo nella consapevolezza che ormai quella sfida è diventata troppo grande per essere affrontata dai singoli anni fa, quando c'erano altri Paesi europei che ritenevano di avere una strategia nazionale e gli interessi del Paese da difendere in Libia? Non ne parlano più, stanno cercando di rivedere la loro presenza nel Sahel e, in un certo senso, di ridurre la presenza per affidarsi di più ad un'azione collettiva e concordata. E qui c'è l'altra evoluzione che, secondo me, è positiva: prima giravamo in ordine sparso, ci danneggiavamo ed eravamo concorrenti; oggi non si parla più di posizioni diverse, ma si discute e si marcia sulla stessa linea.

(dire che blocca ogni riforma è esagerato, perché in fondo di strada ne abbiamo fatta tanta, anche con l'unanimità). Certo che l'Italia si è sempre adoperata perché questo principio fosse superato, ma, siccome per superare il principio dell'unanimità, ci vuole l'unanimità, non ci siamo ancora riusciti.

non solo di gestire l'immigrazione - anche se «gestire» è una brutta parola e preferirei non usarla - ma anche di considerare un aspetto che

perché creiamo potenzialmente nemici della Nazione e del Paese dove devono vivere per forza o per ragione, ma senza poter contare

ci richiama giustamente a fare i compiti a casa, senza aspettare palingenetiche riforme che vengono dall'Europa. Infatti, come ho detto anche prima in risposta al senatore Casini, parecchie cose si stanno facendo e continueremo a farle. Molti interventi hanno toccato il tema dell'atteggiamento e della posizione politica che si deve avere nei confronti di Paesi che presentano aspetti autocratici violazioni dei diritti umani, dei diritti civili e delle libertà politiche, imprigionamenti forzati, utilizzo dei lavoratori come schiavi e così via. Alcuni di questi sono grandi Paesi, per cui, se vogliamo risolvere o comunque affrontare il problema del cambiamento climatico, non lo si può fare senza cooperare con la Cina.

Per questo il ritorno degli Stati Uniti al tavolo multilaterale, coinciso con l'arrivo di Biden, è così importante, perché si è unito alla lotta mondiale per combattere il cambiamento climatico. *(Applausi)*. Con la stessa logica, è molto importante cooperare con la Cina e anche con l'India, che è l'altra fonte

Di questi Paesi, o per un motivo o per l'altro, tutti hanno bisogno per qualcosa. La cooperazione è solo il primo passo. Il secondo - e questo è specialmente vero per la Cina - è la concorrenza. Siamo concorrenti

Quindi ci dobbiamo difendere dalla concorrenza sleale. *(Applausi).* Il terzo pilastro della strategia concerne la posizione che dobbiamo tenere per quel che riguarda, come dicevo prima, i diritti umani, le violazioni della libertà personale, le discriminazioni di ogni tipo. temi bisogna essere franchi. In altre parole, gli accordi e la cooperazione sono importanti, ma altrettanto lo è la franchezza

cooperazione, concorrenza, franchezza e coraggio.

di un altro strumento di un confronto geopolitico che sta avvenendo in tutto il mondo, soprattutto in Africa. Quindi è bene che il G7 abbia preso questa iniziativa.

Mi soffermo un momento sulla discussione in corso in questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione. Ciò che però voglio dire, specialmente rispetto agli ultimi sviluppi, è che il nostro è uno Stato laico

nelle competenti Commissioni parlamentari: è di nuovo il Parlamento che, per primo, discute della costituzionalità. *(Applausi)*. Poi ci sono i controlli successivi della Corte costituzionale. Voglio infine precisare un punto che si ritrova in una sentenza della Corte costituzionale del 1989: la laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ma tutela del pluralismo e delle diversità culturali. Infine, per completare l'informazione, ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all'orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza ovviamente entrare nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il Governo la sta seguendo,

Al senatore Crucioli, che mi ha ricordato giustamente come il bicchiere può essere visto come mezzo pieno o mezzo vuoto, dico che evidentemente lo vede sempre mezzo vuoto,

sono aumentati moltissimo, ma guardi che erano aumentati anche prima del Covid-19; chiaramente sono aumentati anche durante e dopo il Covid. Questo vuol dire che andiamo male? No, vuol dire che ci sono i poveri, che bisogna affrontare la povertà e che, allo stesso tempo, l'economia si sta riprendendo e lo sta facendo bene,

una solidarietà che, nei confronti delle categorie che più beneficiano del reddito di emergenza, spesso si dimentica. Ci sono infatti le categorie che

Caritas: fino a pochi mesi fa, avevamo il fenomeno per cui, per la prima volta nella storia, più del 50 per cento di coloro che stavano nelle file della Caritas era italiano. Speriamo che questo cambi rapidamente, ma non si tratta di ignorare il problema, bensì di vedere che esiste e di riconoscere che la situazione sta migliorando e ci porterà un aiuto anche su quel fronte.

per forza di cose un'epoca di grandi impegni di spesa. Pensate soltanto a quello di cui abbiamo discusso oggi: la pandemia, la cooperazione internazionale, la ripresa economica, i vaccini e le donazioni. Non è il momento di pensare o immaginare un'imminente austerità. Il Patto di stabilità e di crescita, così com'era prima, è superato e questa ormai è convinzione comune. Saranno circa tre anni che continuo a osservare che le regole fiscali che avevamo non erano più adeguate, ma oggi è definitivamente superato. Abbiamo tutto il tempo per una discussione che mi auguro sia equilibrata e informata, perché, sulla base di quanto mi ha detto il commissario Gentiloni,

ancora al senatore Crucioli sulla stagionalità del virus, non c'è alcun dubbio che la situazione vaccinale ed epidemiologica abbia beneficiato della stagionalità,

focolai che si possono creare e ad affrontarli rapidamente. In merito alla continuazione della cooperazione con le Regioni, non rammento chi ricordava che il rapporto tra Governo e Regioni è buono ed è molto importante che resti così.

Questi non hanno finito il loro compito: dobbiamo tenere alta la mobilitazione, perché non sappiamo cosa ci aspetta.

con il senatore Ferro sul fatto che la qualità degli investimenti che facciamo è fondamentale. Dicevo ieri, in occasione della cerimonia del PNRR con la Presidente della Commissione che quello che spero, mi auguro e voglio è che questi soldi siano spesi bene e ciò significa con efficienza, ma con onestà. Quindi la qualità degli investimenti e l'onestà delle nostre procedure e della nostra spesa sono fondamentali per la nostra crescita, ma anche per dimostrare al resto dell'Europa, a Paesi i cui cittadini hanno pagato le tasse per finanziare il nostro PNRR, che questi soldi non sono stati spesi male. Per questo è così importante e la responsabilità che abbiamo è così forte nei confronti di noi stessi e del resto d'Europa.

proprio per riuscire ad arrivare nelle zone lontane subito. Comunque, a parte la telemedicina, il supporto territoriale è molto presente sia nelle politiche attuali, sia nel PNRR. senatore Marco Pellegrini, osservo solo che siamo tutti europei, come ho già detto prima. senatrice Garavini richiama giustamente il fatto che bisogna combattere i fattori che provocano l'immigrazione. Questo è esattamente quello che si intende per dimensione esterna dell'Unione europea, una parte della quale significa

ricordato che c'è stata una discussione tra quelli che volevano sospendere i diritti di proprietà sui brevetti,

La questione si sta avviando verso una strada che definirei costruttiva. La Commissione ha presentato una proposta all'Organizzazione mondiale del commercio

Si stanno nel contempo individuando siti produttivi in Africa, ma non basta, perché, anche qualora si facessero questi due passi, che sono ancora tutti da fare, produrre i vaccini è complicato. Ci vuole trasferimento di *know-how* e, in sostanza, la cooperazione del settore privato, la quale devo dire che nel Global health summit

fatto in tutto due miliardi di dosi, che verranno date all'Africa e ai Paesi a basso reddito al prezzo di costo e ai Paesi di medio reddito con un piccolo profitto. Quindi la discussione è stata estremamente fertile, perché ha portato a un'azione immediata del settore privato e a una proposta della Commissione che si spera possa essere accettata. Al senatore Zaffini, che ricordava i vari problemi dell'Organizzazione mondiale della sanità,

Questo è adesso l'obiettivo principale, proprio in vista di un autunno che non sappiamo come potrà essere. La senatrice Boldrini invita a essere cauti, sempre sul fronte della vaccinazione. Certamente: bisogna apprezzare i miglioramenti, ma non è il momento dei trionfalismi. Non voglio ripetere quello che ho appena detto. È il momento di stare...

Mi sembra di aver risposto a molte domande. Al senatore Lorefice vorrei ricordare che gli immigrati di cui ha parlato sono non 27.000, ma 19.000.

siamo passati da una gestione abbastanza nazionalistica delle posizioni a una condivisa. Come dicevo prima, ci sono Paesi che hanno tassato i cittadini, perché ci potessero dare i *grant* e i sussidi del PNRR.

Chiedo al sottosegretario Amendola di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

Signor Presidente, non userò tutti i cinque minuti a mia disposizione, perché ho già parlato in precedenza. Voglio dire al Presidente del Consiglio che ho apprezzato molto le analitiche risposte che ha dato. Il Parlamento non è un applausometro, non serve per applaudire il Governo,

sono in condominio esattamente tra Governo e Parlamento. A questo proposito, devo dire che su tutto il merito ci possiamo dividere, sul fatto che il Parlamento sia legittimato a esprimere la propria libera opinione e che il nostro sia uno Stato laico in cui c'è distinzione tra le convinzioni religiose

molto distante da noi, da Paesi di altre culture e religioni dove c'è lo Stato teocratico, ma questo non è il nostro Stato. Voglio aggiungere, sul tema della Libia, che mi è chiarissimo, signor Presidente, che lì Italia e Francia - che lei, diplomaticamente, non lo ha citato, ma sa bene che questi sono i problemi - sono andate in ordine sparso. Oggi, purtroppo, rispetto a prima, l'Europa si trova ad agire quando sul campo Russia e Turchia hanno i loro uomini ed è per questo che la Conferenza di Berlino oggi chiede che la data delle elezioni non sia posticipata e che se ne vadano le truppe mercenarie dalla Libia. Evidentemente, dovremo fare di tutto perché queste truppe se ne vadano, affrontando grandissime difficoltà. A nome del Gruppo per le Autonomie, esprimo l'adesione alla proposta di risoluzione di maggioranza, di cui siamo parte convinta.

quello successivo, di ottobre, la vedrà probabilmente ancora al Governo, perché il sistema elettorale tedesco prevede una lunga trattativa prima che si formi un nuovo Esecutivo, ma non vedrà più la Cancelliera nel pieno dei suoi poteri. Parto da questo, signor Presidente - nel ringraziarla e nell'augurarle buon lavoro, assicurandole il sostegno anche del Gruppo Italia Viva

anni di *leadership* merkeliana in Europa solo molto di più di una semplice stagione. Quello di Governo in Germania sarà un cambio di era, non solo un cambio di Governo, sotto questo profilo, è interessante capire quale ruolo potranno giocare l'Italia e il presidente del Consiglio

le ha tributato una *standing ovation* per quello che ha fatto sul ruolo dell'euro e per quello che sta facendo in Consiglio europeo; poi l'incontro con Angela Merkel ed infine a Cinecittà ieri, in un ambiente simbolico e affascinante, quale quello del Teatro 5, l'incontro con Ursula von der Leyen per la presentazione del PNRR, che lei ricordava, signor Presidente, sta cambiando totalmente l'Europa che abbiamo conosciuto solo pochi anni fa, come ricordava anche il presidente Monti.

finiti i tre anni di populismo di questo Paese, l'Italia può tornare ad essere *leader* a livello internazionale e il punto di riferimento anche perché, accanto alla fine dell'esperienza Merkel, ci sono una situazione francese complicata e una battaglia elettorale in Francia resa molto difficile, come abbiamo visto anche nelle elezioni amministrative appena svolte. In questo scenario, ci sono il ritorno prepotente dell'America - «*Diplomacy is back*», come ha detto il presidente Biden qualche giorno fa, dopo il G7 in Cornovaglia - e l'Italia, che è il punto di riferimento del G20, perché quest'anno la Presidenza tocca al nostro la parentesi dello scorso anno, si torna al vertice in presenza a Roma, a novembre. Tutto ciò porta a dire che in questa stagione di due anni che ci separa dalla scadenza naturale del mandato del 2023

Ci sono due Next generation EU. Non c'è soltanto la necessità di intervenire sulla grande e complicata questione dell'emergenza pandemica stando attenti. Condivido il riferimento alla crescita dei contagi anche in quei Paesi dove i vaccinati sono numerosi

scoprire che, a fronte di 127.000 decessi, nel frattempo qualcuno lucrava e rubava sugli approvvigionamenti. Accanto a questa battaglia nazionale che riguarda l'Italia, c'è il ruolo dell'Italia nel mondo c'è il ruolo dell'Italia nel mondo e in Europa. Paradossalmente, per una serie di coincidenze che qualcuno forse aveva intuito, mentre altri non l'avevano fatto, questa è una fase nella quale tra il G20, la *co*-*leadership* della COP26, la fine dell'esperienza Merkel, le difficoltà di campagna elettorale della Francia e la Brexit l'Italia può giocare il ruolo di guida. È chiaro o no che la nostra capacità di sostenere il Governo, oltre naturalmente ai meriti personali del Presidente del Consiglio e della sua squadra, diventa decisiva per dare non all'Italia, ma all'Europa l'orizzonte di cui ha bisogno? Ciò vale, a maggior ragione, per ciò che è stato detto sul Patto di stabilità e sulle regole del bilancio. È vero infatti che sarà nel 2023, ma è nel 2022 che si gioca la partita nei confronti, nei tavoli e nelle discussioni. Ciò vale anche per la grande questione africana,

forse è il momento di dire che sull'immigrazione, visto che in quest'anno possiamo discutere anche con maggiore tranquillità interna, il dibattito va tolto agli *influencer* e va ripreso nella logica della politica.

già vanno all'estero a studiare. Sono migranti diversi da quelli che arrivano a Lampedusa, ma siamo figli e padri di migranti. Essere contro l'immigrazione è come essere contro l'alba o il tramonto. Potete essere contro il fatto che domani mattina spunti l'alba, ma spunterà lo stesso. il problema è come discipliniamo questa grande questione. Ciò che voglio dire è che la questione africana non è soltanto la pandemia né soltanto l'immigrazione; è una questione ben più grave in questa fase ed è legata al ritorno dell'estremismo di matrice islamica. Facciamo attenzione, perché non ne parla nessuno, dico "nostro" perché era uno dei primi Paesi che, anche nella scorsa legislatura, visitammo per tutta una serie di iniziative, di interventi e di investimenti, a cominciare dall'ENI - oggi

non legata semplicemente alla paura, alla preoccupazione e al dibattito da Twitter. Ecco perché penso che serva un protagonismo europeo. europeo. Signor Presidente, penso che nei prossimi due anni ci sarà molto da fare in quest'Europa, che è paradossalmente a rischio, perché il dibattito tra Stati Uniti, da un lato, e Russia e Cina, dall'altro, rischia di schiacciarci e di non farci toccare palla su tutti i grandi temi dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose, dell'innovazione tecnologica, del rilancio di una visione di di medicina personalizzata e di sanità innovativa. L'Europa può avere un senso se noi aiuteremo il nostro Governo a fare ciò che l'Italia deve fare da sempre e che non sempre è stata capace di fare. spesso siamo ripartiti, che è un'isola nel nostro Mediterraneo, il Mare Nostrum. Quanto è importante che lei abbia scelto di fare come prima visita una visita nel Mediterraneo, segnatamente in Libia, anche per evitare mire egemoniche della Turchia, che giustamente contestiamo per il tema dei diritti, ma che dobbiamo contestare anche per una visione sbagliata di geopolitica. Torno in un'isola del Mediterraneo, torno a Ventotene. Era a Ventotene che Altiero Spinelli diceva che la via da percorrere non è facile, né sicura; ma deve essere percorsa e lo sarà. La percorra, signor Presidente; Italia Viva e spero tutto il Parlamento sarà al suo fianco.

Signor Presidente, signor presidente Draghi, sono ore che sente «Grazie, evviva, evviva Draghi!». Ha ricordato molto il fantozziano: «Lei è un bel direttore, un santo, un apostolo!». allora che sarà felice di sentire un coro un po' diverso, con la sincerità e la chiarezza tipica di Fratelli d'Italia. I temi sono moltissimi; ho preparato le *slide* per cercare di stare nei tempi e ho fatto partire il cronometro. Quadro economico positivo: purtroppo non è così, presidente Draghi. Nel 2020 abbiamo avuto un calo del PIL dell'8,9 per cento; la stima Istat per il 2021 è più 4,7 per cento. Si chiama rimbalzo, lei lo sa meglio di me, e vuol dire che la nostra economia è messa malissimo. Abbiamo un milione di posti di lavoro già persi e molti a rischio. L'Istat dice che il 45 per cento delle imprese è a rischio chiusura; questo vuol dire una situazione drammatica. Mi ascolti però, presidente Draghi. Ci dice pure che il lavoro del sostegno dal lato dell'offerta è stato fatto e che adesso tocca sostenere il lato della domanda; ma anche questo non è esatto. Abbiamo avuto nel 2020 un calo del fatturato delle nostre imprese di 350 miliardi. Nel 2020 ci sono stati aiuti per 29 miliardi, cioè l'8 per cento di questa perdita; verranno dati nel 2021, siamo a 42,5 miliardi, una piccola percentuale della perdita. Vuol dire che le nostre imprese sono a rischio chiusura. La priorità rimane sostenere le imprese. Piano nazionale di ripresa e resilienza: è il tempo della verità. Adesso che è partito, smettiamo di dire menzogne. Non lei, ma chi l'ha preceduta ha detto che sarebbero piovuti miliardi su imprese e cittadini e che saremmo stati tutti salvi. Ebbene, adesso che avete avuto il tempo di leggere il PNRR, sapete che non è così. Quei soldi non vanno alle imprese in difficoltà, non vanno ai ristoratori, al turismo, alle palestre; nulla di tutto questo. Servono per una grande svolta *green* e tecnologica, che però cosa comporterà nel breve termine? Visto che vi eravate vantati tutti nella maggioranza di aver letto e capito il PNRR in dodici ore, avrete visto che a pagina 251 il Governo dichiara che, in virtù del PNRR, avremo un peggioramento della bilancia commerciale: aumento delle importazioni e riduzione delle esportazioni. Perché? Perché non siamo campioni del mondo in queste due materie (tecnologia e *green*) e quindi andremo a importare. Da chi? Prevalentemente dalla Cina. Questa è una svolta *green* bizzarra. Per fare la svolta *green* importiamo dalla Cina, che è il Paese che inquina di più al mondo. Sotto questo aspetto il 3 luglio, presidente Draghi,

non producibili le bioplastiche, mettendo in ginocchio le nostre imprese. Visto che Sanchez ha detto che, quando lei parla, la gente la ascolta in Europa, si faccia sentire e dica che il 3 luglio non deve scattare il divieto divieto di produzione di bioplastiche e che le nostre imprese non saranno messe in ginocchio. Se vogliamo salvare il pianeta, visto che l'Europa contribuisce solo per lo 0,6 per cento alle plastiche in mare e che il resto deriva prevalentemente dall'India e dalla Cina, poniamo i dazi di civiltà:

sono calati, perché andiamo verso la bella stagione e con l'arrivo della cattiva stagione rischiamo una nuova ondata. Lo avevamo detto al Governo un anno fa, ma Speranza si è messo a scrivere il libro su come abbiamo sconfitto il Covid e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. ha consegnato al generale Figliuolo le proposte di Fratelli d'Italia su come affrontare la terza ondata. Speriamo che questa volta venga letto questo documento, invece del libro di Speranza. sempre sui numeri, signor Presidente Draghi: se mi ascolta, è importante. Continuiamo infatti ad avere un Governo che smentisce i numeri ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità, degli esperti di Oxford e della comunità scientifica.

dell'Organizzazione mondiale della sanità e di Oxford. Se il Governo ha dei numeri diversi, perché non li fornisce? Non possiamo accettare che il Governo dica che non è così, ma i numeri non vengono dati. minuti e trentasei secondi, dunque mi concentro sull'immigrazione. Questo è l'andamento dell'immigrazione: avevamo 2.300 sbarchi illegali nel 2019 e ora siamo a 19.320, nello stesso periodo.

gran parte del resto è della Spagna. In Spagna funziona così: quando governano i socialisti sbarcano, quando governa la destra no e lo stesso avviene in Italia. In Italia sbarcano solo perché la sinistra immigrazionista comanda in Italia dal 2011 a oggi: questo è l'unico motivo per il quale si sbarca in Italia. *(Applausi)*. Invito i colleghi a stampare la cartina dell'Unione europea, perché può aiutare quando si parla di immigrazione. Dire che l'Italia ha una situazione geografica esposta all'immigrazione, vuol dire non aver mai aperto una cartina geografica. Tutti i Paesi dell'Est Europa hanno confini esterni più esposti dei nostri, perché è più facile attraversare illegalmente il confine dall'Ucraina alla Polonia, che non attraversare il Mediterraneo: non è che ci vuole proprio un genio per capirlo. Anche via mare è più facile arrivare a Malta, in Spagna, a Cipro o in Bulgaria piuttosto che in Italia. Perché sbarcano in Italia? Perché governa la sinistra immigrazionista!

banalmente, come fanno tutti gli altri. Si fa grande polemica perché i cattivoni di Fratelli d'Italia chiedono il blocco navale e l'affondamento delle navi illegali. Lo sapete che questo è quanto chiede l'Unione europea? No, perché non studiate. «l'Unità» del 28 gennaio 2017 pubblica una bella foto della Mogherini: «Unione Europea. Blocco navale in Libia contro le morti in mare». Questa è la soluzione chiesta nel 2017 dalla Commissione europea.

attraverso misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati. Somiglia un po' ad affondare le navi degli scafisti? Sì, e lo chiede l'Europa. Che cosa chiede, invece, la risoluzione di maggioranza? E qui siamo allo scandalo! Volete legalizzare l'attività illegale delle ONG. Al punto 21 della risoluzione di maggioranza c'è scritto: «In modo da assicurare una gestione controllata e legale delle partenze...

sono tempi decisamente nuovi quelli che ci troviamo a vivere e, soprattutto, quelli che siamo chiamati a costruire. Tempi che ci portano, con una sensibilità altrettanto rinnovata, a misurarci con un diverso approccio sui temi, sugli impegni, su prospettive e priorità. Questo mese di giugno, in particolar modo per il nostro Paese, è un mese significativo, che ci riempie di orgoglio, come ha sottolineato lei, presidente Draghi, anche in queste ore. Se, da una parte, giorno dopo giorno, siamo confortati dai dati di monitoraggio della pandemia, che finalmente restituiscono una curva dei contagi che si assottiglia, grazie soprattutto alla sempre più corposa diga dei vaccini, dall'altra parte, sotto il profilo internazionale sono molti i segnali di un vero e proprio risveglio del multilateralismo: con il ritorno della guida democratica alla Casa Bianca, *America is back*, ma, allo stesso tempo, anche con l'Europa che torna ad interpretare un significativo protagonismo interno ed esterno. In questo senso, i temi sul tappeto del prossimo Consiglio europeo sono da considerare come un forte incentivo a continuare a rafforzare il percorso politico dell'Unione. Non c'è dubbio alcuno che la pandemia da Covid-19 abbia rivelato la fragilità dell'euroscetticismo, portando alla luce del sole, sì le debolezze, ma, nel contempo, il senso di comune destino che ci appartiene, come Europa e come europei. Come lei ha detto, oggi fa piacere scoprirci finalmente tutti europei. la questione della vaccinazione diventa elemento centrale, non solo nella strategia di contrasto al Covid-19, ma diventa espressione dell'indirizzo politico che l'Unione intende perseguire e declinare; indirizzo che leggiamo bene nell'impegno per lo sviluppo e la produzione di un accesso equo ed universale ai vaccini anti-Covid-19, non solo in Europa, ma anche nei Paesi del Sud del mondo, quelli più deboli. Il comune destino, che pone non solo l'Europa, ma l'intera umanità di fronte al Covid-19, deve esplicitare, in modo ancora più evidente, quel vincolo di solidarietà umana che la pandemia ha decisamente contribuito a ridestare, quella solidarietà che ha avuto opportunamente modo di declinarsi nell'Unione europea, anche sotto gli aspetti generazionali ed economici, attraverso il Next generation EU ed il nostro PNRR in particolare. Signor Presidente del Consiglio, in questo senso la promozione a pieni voti da parte della Commissione europea del Piano italiano, che riconosce al nostro Paese di aver affrontato le raccomandazioni specifiche ed il rispetto degli obiettivi su transizione climatica e digitale, è un grande successo un grande inizio per il nostro Paese e di questo dobbiamo giustamente restare orgogliosi. Mi permetta quindi di rinnovare in quest'Aula la mia soddisfazione per il lavoro che il Governo ha svolto in questi mesi e al quale il Parlamento tutto ha sinceramente voluto contribuire in termini di osservazioni e proposte, perché abbiamo letto tutti in maniera molto chiara l'importanza e il valore dello strumento messo a disposizione dall'Unione europea. Una svolta

riguardo alla necessità di impegnare i prossimi anni nel totale assorbimento del divario di genere e generazionale che grava in tutto il nostro Paese. modo, condivido pienamente la sua indicazione di riconoscere allo strumento del PNRR la funzione di prima leva per ripristinare una sana equità nel nostro Paese, perché il divario di opportunità, garanzie e diritti esistente tra i diversi territori rende l'Italia meno competitiva e meno pronta ai processi di nuovo sviluppo che il Piano stesso prevede e ci indica, una disomogeneità di diritti che purtroppo, nella maggior parte dei casi, trova - ahimè - una definizione geografica ben precisa, dal momento che nel Mezzogiorno, non solo insiste con maggiore incidenza, va purtroppo a sommare ad ulteriori squilibri, sperequazioni e ritardi atavici che la pandemia ha reso ancora più drammatici. Ne è prova il processo di Build back better, di cui il PNRR è espressione e che per diversi aspetti non può essere esteso al Mezzogiorno, dal momento che non si può ricostruire quello che è sempre mancato. è sempre mancato. Tale situazione, di fatto, rende ancora più stringente l'impegno a introdurre servizi e infrastrutture e a riconoscere diritti universali che non sono ancora oggi presenti e sono effettivamente poco accessibili per i cittadini del Sud. Da questo punto di vista, signor Presidente, la riuscita o meno del PNRR non avrà alibi, non necessiterà di particolari commissioni e di valutazioni *ex post*, dal momento che che sarà plasticamente giudicata da come saremmo stati in grado di migliorare la vita di ogni singolo cittadino, soprattutto nei territori più fragili e per i cittadini del futuro. riprendendo i temi dell'agenda del prossimo Consiglio europeo, riguardo alla questione migratoria occorre che l'Unione continui nella sua lotta contro il vecchio fantasma dell'individualismo, che spesso si è mascherato con un insopportabile sovranismo nazionalista, e ricerchi una soluzione politica, non solo riguardo alla condivisione nella gestione degli arrivi, ma anche alla ricerca di uno strumento capace di instaurare in maniera stabile tavoli autorevoli con gli Stati attori dei movimenti migratori, un impegno che richiede un'attività che coinvolga innanzitutto i nostri *partner* europei, perché è profondamente sbagliato e insostenibile un approccio per così dire *cherry-picking* della partecipazione all'Unione europea. Ci sono oneri e onori che devono essere contemperati e questo va reso chiaro a tutti, anche a chi come la Turchia continua a fare orecchie da mercante sui diritti umani. Anzi, da questo punto di vista aggiungo che il primo elemento su cui intervenire, presidente Draghi, senza sconti, è far riconoscere come superato il Regolamento di Dublino: questo è imprescindibile, altrimenti l'ottimo lavoro fatto dal ministro Lamorgese rischia di non essere sufficiente. Riguardo alla Libia è certo importante e fondamentale il ruolo politico e diplomatico che l'Italia ha recuperato a favore del processo di stabilizzazione per poterlo rimettere in piedi il prima possibile, ma occorre rilanciare un sistema di scambio economico fondamentale per contribuire a normalizzare un territorio dilaniato dal conflitto e dalla presenza di milizie estere che condizionano fortemente la vita di quel Paese. tuttavia ormai incombente e sempre più pressante anche l'impegno per l'Unione a mettere mano a un nuovo assetto istituzionale che superi gli attuali metodi che rallentano l'efficacia dell'azione di Commissione e Parlamento e che trovano giusta sede e occasione di approccio proprio nel prossimo appuntamento della Conferenza sul futuro dell'Europa, che dobbiamo rendere pragmatica e produttiva. Questo assetto, io credo, dovrà comprendere anche gli aspetti legati al bilancio, con la previsione di risorse proprie e di un'unione fiscale, come pure un diverso approccio rispetto alle regole del Patto di stabilità, per accompagnare al meglio i Paesi europei verso l'orizzonte di una ripresa stabile e duratura. Una ripresa che non possiamo limitarci ad ancorare alla conversione al *green* e al digitale, ma che ci chiama a un necessario ulteriore momento di riflessione sulla debolezza strutturale europea sul fronte della ricerca, della sanità e dell'approvvigionamento dei beni e delle materie prime, che la pandemia ha messo in evidenza. Per dare un senso compiuto a questa primavera europea dobbiamo cominciare a costruire anche una nuova strategia industriale di respiro europeo. Siamo infatti alla vigilia di un processo di ripensamento delle politiche della globalizzazione e il recente vertice del G7 in Cornovaglia è espressione anche di una nuova definizione, di un nuovo assetto dei rapporti internazionali, che porteranno ad un maggiore protagonismo dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America, sia sul fronte interno, sia nei rapporti con i Paesi terzi. Concludo, signor Presidente. Una delle tante lezioni che la pandemia ci ha dato è che non possiamo più permetterci di dipendere dai Paesi terzi, Cina *in primis*, per la fornitura di

le ha formulate, la stessa che cercherò di utilizzare io nei pochi minuti che mi sono concessi per fare alcune considerazioni in reazione alla sua relazione, ma anche alla sua replica, oltre che al dibattito che ho ascoltato con grande attenzione. il Consiglio europeo discuterà temi decisivi per l'Europa dei prossimi anni, in uscita da questa crisi; avviene anche a valle di una serie di appuntamenti internazionali, di cui abbiamo discusso anche in questa sede e di cui lei stesso, Presidente, è stato uno dei protagonisti. Penso, appunto, al G7 e al vertice della NATO, in cui è emerso un messaggio molto importante, ossia che quel legame tra l'Europa e gli Stati Uniti, che naturalmente è un legame di natura economica e sul terreno della cooperazione tecnologica e militare, è anche un legame storico e persino sentimentale e oggi si può riaggiornare e rafforzare in ragione del fatto che ci misuriamo con una nuova amministrazione statunitense e con la fine - per fortuna, aggiungo della Presidenza Trump. Tuttavia, Presidente, c'è un compito che spetta a quelle che un tempo venivano chiamate le democrazie occidentali: dimostrare, in questa stagione della storia, che il cosiddetto modello di democrazia liberale è ancora quello che funziona. Infatti, i sistemi che noi chiamiamo non democratici vogliono in qualche modo dimostrare il contrario e l'onere della prova cade esattamente su di noi. Certo, dobbiamo essere molto fermi nei confronti di questi sistemi nel chiedere il pieno rispetto dei diritti umani e civili, gli stessi su cui abbiamo bisogno di avanzare anche nelle nostre democrazie, per esempio, promuovendo leggi di civiltà come quelle contro i crimini d'odio, nel segno del rispetto dell'autonomia del Parlamento e della laicità dello Stato (e ha fatto bene a sottolinearlo). e della laicità dello Stato (e ha fatto bene a sottolinearlo). Ma tutto questo non basta. Infatti, se noi vogliamo dimostrare che le democrazie liberali sono ancora quelle che funzionano, non basta una dichiarazione finale di un vertice internazionale. Occorre, presidente ciò di cui lei stesso ha parlato anche nelle sue repliche, oltre che nella sua relazione, ossia un cambio di passo rispetto ai meccanismi di funzionamento di questi sistemi. La tesi per cui le democrazie liberali non funzionano rischia di fare presa innanzitutto tra le nostre popolazioni e noi a questo dobbiamo reagire, rispondendo, però, con fatti politici, che producano conseguenze anche e soprattutto sul terreno delle condizioni materiali delle persone. Se n'è parlato: noi non possiamo immaginare di uscire da questa crisi ricostruendo i termini di una discussione e l'impianto di quel Patto di stabilità e crescita per come l'abbiamo conosciuto. Ma, come lei stesso ha detto, c'è un convincimento condiviso a livello europeo, ma ci sarà anche una battaglia politica forte da fare. Sulla crescita, le cifre citate (il 4,2 per cento quest'anno e il 4,4 per cento per l'anno prossimo di crescita del prodotto interno lordo) devono farci gioire. Però, presidente Draghi, è importante anche guardare nella scatola nera di questa crescita: ci sono dati che parlano di una crescita che rischia di essere dai piedi dai piedi d'argilla se è trainata, ad esempio, dal lavoro povero, dal lavoro precario, dal lavoro sottopagato. Il tempo determinato è tornato a crescere, così come è tornato a crescere il *part time* involontario: quelle forme che alimentano,

il tema del salario minimo legale dentro la cornice della contrattazione. Occorre anche parlare di cosa è diventata quella catena di appalti e subappalti in cui poi si perde di vista il principio di responsabilità: chi fa che cosa e in capo a chi è la responsabilità dei fatti gravi che accadono in quel meccanismo. Il secondo tema è l'immigrazione. È apprezzabile il superamento di Dublino,

«aiutiamoli a casa loro», ma come principio di un lavoro proattivo dell'Europa nel costruire condizioni di riscatto e di crescita di quel continente. Però dobbiamo dirci anche che esiste immigrazione illegale in questo Paese perché ci sono leggi che l'hanno definita tale; non ci sono infatti possibilità di ingressi legali nel nostro Paese. Questa discussione prima o poi andrà fatta.

l'incontinenza mediatica e verbale di chi, anche dentro questa maggioranza, cerca di mettere un cappello politico su ogni allentamento delle misure di sicurezza. Se oggi possiamo guardare con qualche elemento di speranza la prospettiva davanti a noi è perché c'è stato chi, dentro questa maggioranza e nel Governo, ha tenuto il punto sul principio della tutela della salute pubblica, e noi questo lo dobbiamo riconoscere. Dobbiamo stare su quel terreno, continuare e dirci che la gradualità con cui usciamo da una condizione di emergenza deve essere la cifra dell'iniziativa governativa e parlamentare dei prossimi mesi. Mi avvio C'è un grande capitolo di cui si è discusso ed è quello dei vaccini e quindi anche dei sistemi di protezione intellettuale dei brevetti attorno al meccanismo dei vaccini. Io sono un sostenitore della sospensione dei brevetti lei oggi ci ha detto che la Commissione europea ha indicato una sorta di terza via, che ha definito attribuzione obbligatoria delle licenze. Non ho motivo di pensare che questa via non sia più o meno efficace rispetto alla prima, cioè la sospensione dei brevetti; so però che è un obiettivo da raggiungere nel modo più veloce possibile, perché da questa pandemia usciamo se copriamo in modo velocissimo

di questa consapevolezza si deve dotare e spero, signor Presidente, che almeno a parte di queste osservazioni lei le possa portare autorevolmente in seno al Consiglio europeo. La ringrazio

il prossimo Consiglio europeo giunge dopo due appuntamenti internazionali di rilievo quali i vertici G7 e NATO, che hanno evidenziato una significativa comunione di intenti tra i principali *partner* globali, pur con alcuni distinguo interni all'Europa; accenti e sensibilità che riguardano anche temi all'ordine del giorno del Consiglio e che pertanto necessitano da parte nostra di un approccio pragmatico, consapevole, non retorico, in linea con in linea con quanto lei ha fatto in questi primi mesi di vita dell'Esecutivo. Tra questi temi è evidente che il *dossier* economico e il *dossier* migranti hanno una rilevanza particolare, pur personalmente considerando fondamentale per la necessaria protezione internazionale del nostro Paese, specie sul versante Mediterraneo, la sempre più rilevante questione turca e il tema dei rapporti con la Russia. I Paesi europei, nonostante alcuni errori non secondari, stanno procedendo verso una vaccinazione di larghi strati della popolazione. Serve proseguire su questa strada, garantire forniture vaste e crescenti di vaccini agli Stati, non solo quelli europei, ma cominciando da quelli limitrofi, e predisporre un'azione comunitaria per il futuro, per far fronte eventualmente all'insorgere di recrudescenze. Presidente del Consiglio, crediamo si debbano riaprire definitivamente i confini e sapere che in autunno, anche innanzi ad aumenti dei contagi, dovremo imparare a convivere con un virus che diventerà endemico. Se sul fronte economico registriamo i primi risultati positivi con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nonostante le sollecitazioni provenienti da un'istituzione a lei cara come la Banca che sottolinea la necessità che l'economia sia sostenuta da adeguati stimoli sia monetari sia fiscali, si intravedono all'orizzonte i rischi di un rigurgito rigorista, di politiche di *austerity* fuori dal tempo e dalla storia a cui certi Paesi membri e alcune realtà interne a loro guardano con simpatia. È una discussione che forse è sfuggita a molti, ma non certo a lei, signor Presidente del Consiglio, anche perché alcuni suoi teorici, come l'ex ministro tedesco Wolfgang Schäuble, oggi presidente del Bundestag, la chiamano in causa, nel mentre sostengono, prima dalle colonne de «Il Sole 24 Ore» e più di recente da quelle del «Financial Times», la necessità di ripristinare al più presto una severa disciplina fiscale. Sono parole che fanno il paio con le dichiarazioni non smentite del commissario Dombrovskis, che poche settimane fa ha parlato del ripristino del Patto di stabilità nel 2023. Signor Presidente del Consiglio, lei ha detto che abbiamo tempo e ha speso parole di ottimismo e di certo non possiamo e non dobbiamo dare a lei suggerimenti e consigli su questa materia; però che tutti noi, tutto il Parlamento debba essere ben consapevole che in seno all'Europa la battaglia contro il rigore non è finita e che da essa dipendono il nostro futuro e gli spazi di libertà, di sovranità e di agibilità democratica del nostro Paese, nonché i destini della stessa Unione europea, che necessita sempre più di una grande riforma, di una nuova stagione costituente che metta la parola fine a totem e feticci che l'hanno portata da affrontare impreparata sfide che sono state epocali. Su questo le chiediamo un impegno forte, consapevoli che la sua autorevolezza può rappresentare un valore aggiunto, una forza per impedire nel prossimo futuro un pericoloso ritorno al passato. Mentre dobbiamo evitare pericolose fughe all'indietro, abbiamo la necessità, ormai davvero inderogabile, di andare avanti sul *dossier* migranti. Presidente del Consiglio, senza mezzi termini, ma con responsabilità e senza dogmatismi diciamo che le proposte contenute nel nuovo patto europeo per l'immigrazione e l'asilo non sono minimamente soddisfacenti per l'Italia. L'impianto complessivo non affronta risolutivamente il problema che poniamo come Paese. Manca un effettivo meccanismo di solidarietà e ripartizione dei migranti, che necessita di un sistema di accoglienza europeo che porti ad un ricollocamento automatico fra tutti i Paesi dell'Unione *(Applausi)*. Un meccanismo obbligatorio che preveda sanzioni. La dimensione europea dei confini è la giusta prospettiva, come è giusta l'idea di sviluppare intese comunitarie con il Nord Africa, essendo sostenuti in questo anche dall'interesse tedesco di vedere rinnovate le risorse date ad Ankara. Prospettiva a cui aggiungerei la suggestione di allargare all'area MED gli stessi fondi dei progetti europei per un effettivo partenariato di sviluppo condiviso. Mi chiedo però, e le chiedo, cosa faremo se l'interpretazione in seno al Consiglio sarà più simile a «*mare nostrum*» che non ad un meccanismo di solidarietà? La scelta mediterranea, che deve essere la scelta prima dell'Europa e dell'Italia, necessaria per chi vuole oggi svolgere un ruolo non marginale nella nuova configurazione politica ed economica dello scenario internazionale, ci pone anche dinnanzi al tema dei rapporti in questa area strategica, in cui la presenza russa e turca non sono più secondarie. Peraltro, una tale posizione europea - e coloro che ne sono portatori può produrre, come auspichiamo, un'intesa privilegiata con l'alleato americano, distratto giustamente dal confronto epocale con Pechino, i cui inviti a partecipare alla «Via della seta» non dovrebbero interessarci poiché in netto conflitto con la nostra collocazione atlantica. Per questo credo che il Consiglio, così come provano a fare gli Stati Uniti, debba fare uno sforzo verso la Russia ed evitare di consegnarla, se ancora possibile, definitivamente nelle braccia di Pechino, che rappresenta la vera sfida dell'Occidente tutto e dell'Europa. Ciò non vuol dire mantenere un atteggiamento di indifferenza e di passività rispetto a questioni fondamentali, ma significa affrontare il tema di un partenariato tra Russia e Unione europea, significa ad esempio spiegare che la NATO resta e resterà un'alleanza strategica per le realtà europee, significa anche dire che è impensabile sostenere il regime bielorusso, che soffoca la dissidenza filo-occidentale, che chiede libertà e democrazia. Ebbene, se l'Unione vuole avviare questo dialogo, che io reputo positivo, è necessario anche contrastare gli attacchi russi agli interessi dell'Unione europea, è necessario che l'Unione diventi più robusta e resiliente, come ha detto Borrell, meno divisa, meno opportunista e meno influenzabile. Capiamo bene l'interesse preminente delle realtà mitteleuropee di mantenere chiuso il rubinetto della rotta balcanica finanziando Ankara, ma la Turchia,

specie dopo la recente guerra tra Hamas e Israele. Se Erdogan pensa che la Turchia ha fatto più che abbastanza per consentire a Bruxelles di avviare un'agenda positiva con Ankara, noi pensiamo che qualcosa in più vada fatto soprattutto sul fronte delle questioni regionali - penso alla Libia - e aggiungo sul piano dei diritti umani. Presidente, sappiamo che i nostri timori e le nostre speranze sul piano europeo ed internazionale sono da lei largamente condivise e sappiamo che nonostante alcune scivolate di settori della maggioranza la collocazione internazionale dell'Italia è chiara e salda. Per questo votiamo a favore della mozione di maggioranza,

il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà favorevolmente alla risoluzione n. 2, che porta la firma dei senatori Lorefice, Candiani, Giammanco e altri,

l'impegno al Governo non è solo volto a rafforzare la strategia europea sui vaccini garantendo una distribuzione di carattere universale, ma a potenziare la ricerca per trovare una cura appropriata.

di una puntura una volta l'anno o ogni sei mesi, così come sembra, per tutto il resto della nostra vita. Allo stesso modo, non possiamo pensare che il *green pass,* oggi strumento utile per rilanciare il turismo e la nostra economia, possa diventare in futuro uno strumento definitivo, a sistema, magari nelle mani di uno statalismo terapeutico

Presidente Draghi, ci rassicuri perché la Lega sarà sempre in prima linea nella difesa delle libertà costituzionali.

Draghi, lei ha dichiarato in più di un'occasione che finché la pandemia infuria, il virus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione di maggior successo.

questo è il tema vero - di recuperare il tracciamento (come ha detto in più di un'occasione il sottosegretario Sileri, oggi presente in Aula); la sterilizzazione immediata dei focolai, come ha ricordato bene lei;

finalmente nel Consiglio europeo, oltre a parlare di immigrazione - già questa è una notizia - non si parlerà solo dei ricollocamenti o della ridistribuzione obbligatoria, che è stato un punto che ha visto l'Europa fallire negli ultimi dieci anni, di cui si è parlato per tanto tempo, ma finalmente si parlerà di finanziamenti europei attraverso un incremento di programmi e di progetti di cooperazione

Certo che la strada può essere quella, perché portare investimenti, civiltà, istruzione e sviluppo, anziché presunte missioni di pace, può davvero aiutare la fascia centrale del continente africano, che è l'origine degli importanti flussi migratori e contribuire anche alla stabilizzazione della Libia, come ha detto lei. Disincentivare le partenze, signor Presidente: questo è davvero il tema. Lo dico a tutta l'Assemblea, anche al senatore Renzi, che ha detto giustamente che su questo tema dell'immigrazione si può parlare adesso anche in maniera più tranquilla rispetto al passato, ma lo si può fare anche perché ci sono due *leader*, a livello mondiale, la Prima Ministra danese e la Vice Presidente degli Stati Uniti, che hanno invitato - una attraverso una legge (la Ministra danese) e l'altra attraverso dichiarazioni molto importanti molto importanti - gli aspiranti migranti a restare nella propria patria. Questa è una vera e propria svolta mondiale della sinistra. quindi, potremo affrontare questo tema con pragmatismo e non più con l'ideologia che ci caratterizzava prima,

gentili senatori e senatrici l'Italia arriva a questo Consiglio europeo con la storica notizia dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte della Commissione von der Leyen. È quindi ufficialmente aperta la strada dell'erogazione della prima *tranche* di finanziamenti del Next generation EU, 25 miliardi di euro che arriveranno nel giro di poche settimane e saranno finanziamenti ricavati attraverso l'emissione di debito comune europeo, i famosi eurobond di cui il MoVimento 5 Stelle parla da più di dieci anni e che la settimana scorsa hanno avuto il loro debutto nei mercati finanziari, con un'asta da 20 miliardi, titoli che sono andati letteralmente a ruba. In questi casi, la riflessione sorge spontanea, presidente Draghi:

*(Applausi)*. Sono passati poco più di dodici mesi, ma sembrano decenni per la grandezza della portata innovativa di questo radicale mutamento paradigmatico.

il MoVimento 5 Stelle ha dimostrato in questi due anni come dietro questa parola ci sia lavoro e ci siano le imprese; ha dimostrato come dietro questa parola ci sia il superbonus del 110 Dietro questa parola c'è il Rigenera Italia, una misura per la riqualificazione degli edifici pubblici; dietro questa parola c'è il Proteggi Italia, a contrasto del rischio idrogeologico del territorio italiano; dietro questa parola c'è il disegno di legge "salva mare", cha aspetta solo una spinta di coraggio da parte di tutti voi perché possa vedere finalmente anche il mare un bene tutelato dalla Repubblica italiana.

Josep Borrell, ha spiegato come questo risultato che oggi stiamo festeggiando tutti non era affatto scontato. È stato raggiunto - cito testualmente ciò che lui ha dichiarato - grazie all'atteggiamento combattivo e alla determinazione mostrata dai primi ministri Giuseppe Conte e Pedro Sanchez, grazie agli argomenti solidamente esposti da Italia e Spagna. Borrell ha praticamente detto che tutti noi,

a Giuseppe Conte per il ruolo cruciale che ha svolto per la nascita di questo straordinario strumento economico europeo. è solo l'inizio di una lunga battaglia che il MoVimento 5 Stelle di Giuseppe Conte porterà avanti per continuare a riformare radicalmente l'Europa, per chiudere definitivamente l'epoca dell'*austerity*, per conseguire definitivamente la revisione radicale del Patto di stabilità, per la predisposizione finalmente di un bilancio europeo alimentato da risorse proprie che non pesino sui bilanci nazionali, a partire dalla tassazione delle multinazionali e dei colossi dell'economia digitale. dalla parte dei più deboli. Tralascio le prossime battaglie per l'adozione di nuove regole europee per il contrasto del *dumping* salariale e fiscale che c'è in Europa, per l'introduzione del salario minimo europeo e per la lotta ai paradisi fiscali europei. Non potremo mai parlare di Europa seriamente se non abbattiamo i paradisi fiscali Presidente, lei al Consiglio avrà poi modo di discutere dell'enorme sforzo internazionale volto a garantire un accesso universale ed equo ai vaccini anti-Covid, quindi a vantaggio anche dei Paesi poveri, anche al fine di evitare il proliferare di quelle pericolose varianti (vedo qui il sottosegretario Sileri), che, come dimostra il caso del Regno Unito, mettono a repentaglio addirittura la copertura vaccinale dei Paesi ricchi. Siamo tutti legati, ricchi e poveri, davanti a questa emergenza e su questo il MoVimento 5 Stelle è in prima linea. Ed è per questo che, negli impegni della proposta di risoluzione di maggioranza che ci apprestiamo ad approvare, chiediamo che lo sia anche il nostro Governo, che lo sia anche il Governo italiano, adoperandosi presso tutte le sedi affinché si possa arrivare a una sospensione temporanea dei brevetti e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale. Lo dobbiamo fare, se vogliamo salvarci tutti. su richiesta del Governo italiano (come giustamente lei ci ha ricordato), è stato inserito anche lo spinoso tema dell'immigrazione, che accende ancora la destra sovranista (l'abbiamo visto adesso); tema che l'Italia, fin dal primo Governo Conte, ha posto in maniera rilevante all'attenzione dell'Europa. Ricorderete tutti ciò che accadde nel giugno 2018, quando Conte pose il veto italiano alle conclusioni del Consiglio europeo, riuscendo a portare tutta l'Unione europea a compiere quel primo passo verso un approccio solidale e condiviso. Oggi noi non siamo davanti allo stato di emergenza di quei giorni; tuttavia non possiamo negare che si tratta di un fenomeno che l'Italia fatica a gestire pienamente e compiutamente, perché perché l'Italia è stata lasciata sola, signor Presidente. I numeri sarebbero perfettamente gestibili per un'Unione di 27 Paesi che conta mezzo miliardo di abitanti, in Europa prevalesse quel principio di solidarietà e di condivisione della responsabilità, attraverso l'introduzione di un meccanismo di redistribuzione automatico e obbligatorio di tutti i migranti. Potrei andare avanti, ma vedo che il tempo sta per scadere. Signor Presidente, le posizioni del MoVimento 5 Stelle, su questi e altri importanti temi che saranno discussi al Consiglio europeo, trovano pieno riscontro negli impegni al Governo contenuti nella proposta di risoluzione di maggioranza, che quindi sosterremo con il nostro convinto voto favorevole.

Questo piano è una finzione degna di Cinecittà: la pioggia di soldi è un effetto speciale, la ripresa e la resilienza sono la sceneggiatura che incanta, commuove, fa sperare, almeno fino ai titoli di coda, quando poi scorrere la scritta: «I fatti e i personaggi di questo film sono frutto di pura fantasia». Allora poi bisogna fare i conti con la realtà, che è una: l'Italia sarà commissariata e lei è il commissario perfetto. Altro che ingerenze del Vaticano, qui siamo alla svendita dell'Italia e degli italiani a favore di finanza e multinazionali. Per esempio nel PNRR, a pagina 57, abrogate (precedentemente si parlava solo di una proposta di abrogazione) le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva. In poche parole, state condannando migliaia di famiglie a lasciare la casa prima dell'asta immobiliare; un mutuo diventa una condanna alla disperazione. La legislatura cominciò ridando dignità ai tanti bramini d'Italia. Oggi gliela state togliendo, aggravando la situazione e truffando il Parlamento. Eccola la vostra dimensione sociale: siete avvitati alle più cannibalesche pratiche finanziarie. Ecco dove Federico Caffè vi avrebbe inchiodati alla definizione di «incappucciati della finanza». State sbattendo fuori casa famiglie e piccoli imprenditori, colpevoli di non riuscire a far fronte a un mutuo, nel pieno dell'emergenza Covid. Li vaccinate, ma li fate morire di disperazione. Lo sguardo di Draghi sulla società è diabolico. Il vostro nuovo umanesimo è lo stesso di cui parlava Al Pacino nel film «L'avvocato del diavolo». Vi riempite la bocca di riconversione all'elettrico, ma è solo una grande abbuffata. Arrivano i soldi per il *green*? Evviva! Allora finalmente le bollette saranno drasticamente tagliate, perché gli oneri di sistema saranno completamente a vostro carico e non avrete più scuse. Per il lavoro? Finalmente abbatterete le tasse, non che i *rider* possono essere sfruttati a norma di legge, mentre qui un collaboratore cameriere costa quasi due volte di più rispetto alle multinazionali. Con i soldi dell'Europa pagherete i debiti della pubblica amministrazione, presidente Draghi, o almeno compenserete, una volta per sempre, con gli imprenditori creditori? Oppure sarà la solita partita di giro, sempre a vantaggio della pubblica amministrazione, con l'Agenzia delle entrate nella parte dello sceriffo di Nottingham? Forse vi siete calati troppo nella parte di Harry Potter e i soldi compaiono e scompaiono per magia: ai Benetton sì e ai piccoli imprenditori no. È dal 16 giugno che un pezzo d'Italia aspetta i vostri soldi. Dopo «Totòtruffa» torniamo ai pacchi di Nanni Loy. Stavolta però la regia è sua.

In materia economica, ritiene che io veda sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il punto però non è questo, ma è che non tollero che quel bicchiere se lo bevano sempre gli stessi. Le ho chiesto un intervento specifico, ovvero di prorogare il blocco dei licenziamenti, ma su questo non ha dato alcuna risposta e ha dribblato l'argomento. Allo stesso modo, in materia di pandemia e di vaccini, le ho chiesto delle questioni specifiche, ovvero di adoperarsi per la divulgazione dei dati grezzi, disaggregati, non elaborati e che, ad esempio, sui dati relativi ai nuovi contagiati e ai nuovi deceduti sia indicato quale percentuale di loro avevano già ricevuto il vaccino. È un dato facile da ottenersi e rilevante per fare le valutazioni. Su questo, di nuovo, non ha detto nulla. adottare i protocolli per le cure territoriali che non siano semplicemente tachipirina e vigile attesa e di riconoscere che la vaccinazione sui minori non solo non è una priorità, come ha detto lei, ma è un errore *(Applausi)*, perché i minori non corrono rischi di conseguenze gravi da Covid, ma potrebbero avere degli effetti negativi sia di breve termine - rari, ma ci sono - che di medio o lungo termine, visto che gli studi non sono stati portati a termine. per quanto riguarda il *pass* vaccinale, vada per cortesia in Europa a sostenere che le discriminazioni che si introdurranno con questo *pass* vengano ridotte, ad esempio rendendo gratuiti i tamponi e i test antigenici, per consentire che anche coloro che non si vaccinano, perché non è obbligatorio, possano muoversi in sicurezza, senza correre il rischio di contagiare nessuno. Abbiamo proposto un emendamento per la gratuità di questi test, ma è stato respinto dalla